L'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ne prevede la presentazione alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti, articolandoli in tre sezioni e una serie di allegati. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del Piano di stabilità e crescita. La seconda sezione riporta l'analisi e le previsioni dei dati di finanza pubblica a legislazione vigente, nonché le previsioni a politiche invariate per i principali aggregati. La terza sezione, infine, espone il Programma nazionale di riforma. Dopo l'esame parlamentare, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Il DEF 2024 presenta una struttura più sintetica rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza, in considerazione dell'attuale fase di transizione verso le nuove regole della *governance* economica europea e quindi della predisposizione di un quadro programmatico coerente con le nuove regole europee. Il Governo ha quindi annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo. L'Italia dovrà presentare entro il prossimo 20 settembre il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine, tenendo conto della predisposizione, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento dell'andamento dell'indice della spesa primaria netta. Il Governo si è limitato a illustrare nel DEF 2024 i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica, con una stima delle politiche invariate per il prossimo triennio. Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF 2024 espone l'analisi relativa all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica e di politica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del Documento stesso. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare del bilancio il 10 aprile di quest'anno. Richiamando le stime ufficiali dell'Istat, il Documento evidenzia come il PIL nel 2023 sia cresciuto dello 0,9 per di crescita in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro, che era +0,4 per cento. Il DEF sottolinea che il PIL reale è aumentato di 4,2 punti percentuali rispetto al livello pre-Covid registrato nel quarto trimestre del 2019. Nel complesso, quindi, la crescita nel 2023 è stata trainata dalla domanda interna (4,6 punti percentuali), unitamente alla ripresa della domanda estera netta. La crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico programmatico della NADEF, che era pari a +1,2 per cento, legata - e questo lo si spiega nel DEF - ad una scelta prudenziale, dato l'elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale e il protrarsi di tensioni geopolitiche. L'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe principalmente guidata, secondo il DEF, dall'incremento della domanda interna, sostenuta principalmente dal rientro dell'inflazione e da un allentamento graduale delle condizioni monetarie e del costo del credito. Guardando all'intero periodo previsivo, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 più sostenuta rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 Il DEF sottolinea peraltro che sulle nuove previsioni di crescita, per motivi prudenziali, non è stato considerato appieno lo stimolo fornito dal PNRR e i suoi effetti espansivi dal lato dell'offerta e sulle stime di prodotto potenziale. Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, i dati riferiti al 2023 attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari a 149,5 miliardi di euro, corrispondenti al 7,2 per Per quanto attiene al confronto con le precedenti stime per il medesimo anno, si evidenzia che la NADEF 2023 aveva previsto, in termini di PIL, un indebitamento netto pari al 5,2 per cento su base tendenziale e al 5,3 per cento su base programmatica. Tale scostamento, pari a circa 40 miliardi di euro, con riferimento sia all'indebitamento netto sia al saldo primario, è attribuibile in larga misura all'andamento più elevato delle spese in conto capitale. A fronte infatti di un saldo corrente con segno positivo (+0,6 per cento del PIL) e migliore rispetto alle attese per circa 14,4 miliardi di euro, l'aumento dell'indebitamento netto rispetto alle previsioni è dovuto in particolare ai maggiori contributi agli investimenti per circa 47 miliardi di euro, voce che comprende i contributi riconosciuti nell'ambito della misura cosiddetta superbonus. Per quanto attiene, invece, al confronto con l'esercizio precedente, il dato evidenzia un miglioramento rispetto all'anno 2022. La riduzione del *deficit* dal 2022 al 2023, pari a circa 18,5 miliardi di euro, è dovuta al miglioramento del saldo corrente di circa 35,7 miliardi rispetto all'anno precedente, in parte assorbito da un deterioramento del saldo tra spese e entrate in conto capitale per circa 17,2 Il miglioramento dell'indebitamento netto rispetto al 2022 si riflette anche in un saldo primario tra entrate e spese, al netto degli interessi passivi, che, migliorando di circa 14,2 miliardi di euro, inverte il suo segno, attestandosi su valori positivi. Nel dettaglio, come evidenziato dal comunicato Istat di marzo, le entrate correnti hanno registrato un aumento del attestandosi al 46,6 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono cresciute del 10,2 per cento, principalmente per l'aumento dell'Irpef e dell'Ires; sono in aumento anche le sostitutive sugli interessi e sui redditi

un aumento delle entrate tributarie di circa 15 miliardi. In particolare, le imposte dirette aumentano di 10.807 milioni di euro e le imposte indirette di 4.171 milioni, mentre sono sostanzialmente in linea con le previsioni le imposte in conto capitale: -14 milioni. In proposito, il Documento precisa che, con riguardo ai singoli aggregati (bilancio dello Stato, poste correttive ed enti territoriali) e alle principali categorie economiche, presentano uno scostamento positivo rispetto a quanto previsto le voci classificate nel bilancio dello Stato (+6.716 milioni) Le poste correttive che nettizzano le entrate tributarie sono risultate pari a -34.730 -34.730 milioni, inferiori alle attese, determinando un effetto positivo di 6.975 milioni. Nel dettaglio a consuntivo, il miglioramento delle entrate del bilancio dello Stato è ascrivibile al maggior gettito registrato dalle imposte dirette per effetto, in particolare, dei maggiori introiti delle imposte versate in autoliquidazione Irpef ed Ires. Lo scostamento positivo relativo alle voci delle poste correttive risulta ascrivibile, per 4,5 miliardi, alle maggiori entrate derivanti dalle attività di accertamento e controllo rispetto a quanto previsto. Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali, che hanno fatto registrare nel 2023 un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2022. Le imposte in conto capitale, risultate pari a 1.608 milioni nel 2023, registrano una riduzione di 99 milioni rispetto al 2022. La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,5 per cento, invariata rispetto all'anno precedente, per effetto, come precisato dall'Istat, di una crescita del PIL a prezzi correnti per cento), pari a quella delle entrate fiscali e contributive. In conseguenza dei descritti andamenti, la pressione fiscale rimane sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di previsione:

La variazione complessiva è dovuta essenzialmente alla riduzione dell'incidenza sul PIL della spesa corrente primaria e della spesa per interessi. Tale riduzione risulta parzialmente compensata dall'incremento dell'incidenza della spesa in conto capitale, che passa dall'8,3 per cento del 2022 Nel 2023, la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata pari a circa 424 milioni di euro, corrispondente al 20,4 del PIL, in diminuzione rispetto al rapporto registrato nel 2022. La voce di consuntivo per l'anno 2023 di altre uscite correnti registra una lieve diminuzione di sei milioni rispetto all'anno precedente, con un livello di spesa pari a 96 miliardi

La spesa in conto capitale nel 2023 è risultata pari, in valore assoluto, a 186 miliardi, con un incremento rispetto al 2022 del 14,8 per cento, pari in valore assoluto a 24 miliardi. Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente, il DEF espone l'andamento previsto dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel periodo 2024-2027, sulla base delle informazioni relative al consuntivo diffuse dall'Istat, dall'Istat, del nuovo quadro macroeconomico rappresentato dalla sezione I del DEF medesimo e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2024. Il DEF specifica, in aggiunta, che l'aggiornamento delle previsioni del conto della pubblica amministrazione include anche l'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziate da sovvenzioni a fondo perduto e prestiti nell'ambito del PNRR, alla luce delle modifiche al Piano, approvato dal Consiglio Consiglio dell'8 dicembre 2023. Il Documento di economia e finanza stima un andamento crescente delle entrate finali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del del quale l'aggregato passa da 1.011,6 miliardi nel 2024 a 1.094 miliardi nel 2027. Per quanto riguarda le spese in valore assoluto, i dati stimati per gli anni dal 2024 al 2027 sono pari a pari a 1,105 miliardi. Rispetto all'esercizio precedente, l'aggregato mostra una riduzione nel 2024. Le raccomandazioni specifiche per il 2024, approvate dall'Ecofin e dal Consiglio europeo nello scorso giugno, suggerivano agli Stati membri di impostare le programmazioni di bilancio di medio periodo in modo coerente con i criteri che avrebbero ispirato la riforma della *governance* finanziaria. Il Documento sottolinea come l'indicatore di riferimento per la sorveglianza di bilancio di quest'anno sia la spesa finanziata a livello nazionale, al netto delle spese per per interessi, delle spese relative ai programmi dell'Unione interamente coperte dai trasferimenti provenienti dall'Unione europea, della componente ciclica della spesa per le indennità di disoccupazione, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e delle misure *una tantum* e temporanee. In base all'aggiornamento delle previsioni del DEF in esame nel 2024, l'andamento della spesa primaria netta e l'andamento del saldo di bilancio strutturale del quadro tendenziale possono ritenersi conformi alle raccomandazioni specifiche proposte dalla Commissione europea e approvate dall'Ecofin nel nel 2023 e poi dal Consiglio europeo nel giugno 2023. La tendenza al miglioramento dei saldi strutturali è confermata anche negli anni seguenti. Per quanto riguarda il debito pubblico per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito-PIL in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la dinamica del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL, il DEF evidenzia che i crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al pari degli altri incentivi fiscali, incidono Nel DEF il Governo riporta una stima dell'impatto macroeconomico delle spese delle principali riforme previste previste dal PNRR che tiene conto della revisione del Piano approvato dal Consiglio dell'Unione europea a dicembre 2023. Inoltre, coerentemente con l'approccio adottato precedentemente, al fine di isolare unicamente l'impatto addizionale sull'economia, la valutazione è stata effettuata considerando tra tutte le risorse citate solo quelle che finanziano progetti che possono essere considerati aggiuntivi. Nel DEF il Governo riporta anche un aggiornamento della stima dell'impatto macroeconomico delle principali riforme previste dal PNRR, in particolare quelle relative a istruzione, ricerca, politiche attive del mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti. Il Documento conferma l'elenco dei disegni di legge da qualificare come collegati definito dalla Nota di aggiornamento al DEF 2023. Riguardo all'elenco in precedenza definito, si ricorda la previsione di un disegno di legge recante misure a sostegno delle politiche per il lavoro, di un disegno di legge recante interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà, di un disegno di legge recante interventi in materia di disciplina pensionistica, di un disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale universale (delega al Governo per il riordino della materia) e di un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. La Commissione bilancio mi ha conferito mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame.

si veniva in Aula o si finiva sui giornali ad annunciare grandi progetti di riforma e di innovazione nella politica economica italiana. Purtroppo questo DEF ci

Lo dico perché siamo di fronte a un Documento che non presenta il quadro programmatico, quindi non sapremo esattamente qual è l'indicazione del Governo e come si vogliono gestire le risorse pubbliche nei prossimi anni, né dal punto di vista della spesa corrente, né dal punto di vista degli investimenti. anche in una navigazione al buio, perché i numeri su cui stiamo lavorando sono già stati superati dalla realtà dei fatti. Infatti, proprio mentre discutevamo del DEF, ci sono arrivati gli ultimi calcoli dell'Istituto di statistica,

nel Documento che stiamo approvando, perché si tratta di un inedito. Ora, per chi non si trova a gestire spesso i documenti di economia e finanza, soprattutto quelli così importanti, potrebbero sembrare dati non così indicativi. In realtà questo ci dice che c'è una confusione generale, che non potrà non potrà altro che portarci a una manovra di bilancio che si preannuncia estremamente difficile (non solo quella di quest'anno, ma anche quelle dei prossimi anni). La manovra parte, secondo i calcoli che ci sono stati forniti dall'UPB, con un'incognita di almeno 20 miliardi per coprire le spese temporanee previste nella scorsa legge di bilancio. Lo abbiamo detto anche l'anno scorso: mettere il taglio del cuneo fiscale e continuare a insistere su misure temporanee e non strutturali nella nostra organizzazione mette in pericolo non solo le risorse per i cittadini e i lavoratori, in questo caso, ma anche la programmazione e la visione rispetto alle politiche salariali e alle politiche di attrattività del lavoro nel nostro Paese. In quei 20 miliardi c'è un po' di tutto: le

Non è un caso se ieri, nel Consiglio dei ministri, è stata stoppata la misura sulla tredicesima. Leo è dovuto tornare indietro su una misura importante che era stata annunciata dal Governo con grande enfasi. Vedremo che cosa accadrà sulla delega fiscale, perché il DEF, rispetto anche al nuovo Patto di stabilità, ci chiede almeno lo 0,5 per cento del PIL l'anno, a cui poi si devono aggiungere tutte le altre spese di cui

il debito costa e che questo costo sottrae risorse a cose più importanti, come sanità e istruzione. Infatti, se andiamo a vedere la previsione di spesa per la sanità nei prossimi anni, abbiamo il 6,4 per cento nel 2024 (ma soltanto in virtù del trascinamento dei contratti, in quanto le risorse che avevamo messo da parte e che dovevano essere spese lo scorso anno verranno spese il prossimo),

Sotto il 6,6 per cento non siamo andati neanche durante gli anni della più grande crisi che abbiamo attraversato in Italia, con i famosi tagli lineari. Questa cifra comporta una compressione ulteriore dei servizi sanitari e alla persona nelle Regioni italiane che, oltre

nello stesso DEF e in tutte le audizioni svolte in questi giorni si dice una cosa: l'unico modo che abbiamo per attenuare questa crisi è crescere, far aumentare la nostra produttività

da qui al 2027, è tenuta in piedi dalla nostra capacità di spendere 200 miliardi di euro (occasione che non avremo più) in investimenti per risolvere le diseguaglianze, ammodernare il nostro Paese e dargli una spinta economica rispetto ai numeri desolanti

perché nella condizione di nuova crisi in cui ci stiamo avviando c'è bisogno di una chiamata di tutti noi ad una responsabilità condivisa delle azioni e degli strumenti che verranno messi in campo nei prossimi anni in Italia, per non dover poi piangere per le prossime due generazioni.

Ebbene, stiamo avendo degli indicatori positivi e rilevanti, come per esempio l'inattesa crescita dello 0,9 che abbiamo riscontrato nonostante il 2023, a livello geopolitico, sia da considerarsi l'anno con il maggior numero di conflitti della storia dalla Seconda guerra mondiale ad oggi.

organismi deputati a compartecipare, a commentare e a collaborare nella stesura di documenti così rilevanti. richiamavano l'attenzione su quelle che possono essere, per esempio, anche le strozzature commerciali che adesso stiamo vivendo. Pensiamo allo Stretto di Suez, pensiamo al fatto che l'Italia si è posta alla guida dell'operazione di difesa Aspides nel Mar Rosso per consentire di far arrivare le merci all'Italia. Quello che sto cercando di dire

bilancio della Camera dei deputati, abbiamo dato degli indirizzi chiari al nostro Ministro e al nostro Governo per portare avanti questo difficile negoziato con l'Unione europea

dato una serie di indirizzi chiari, quali ad esempio il fatto che fosse previsto che il Piano strutturale di bilancio a medio termine privilegiasse in modo riscontrabile ed eventualmente apportando trasparenti modifiche un approccio favorevole alla crescita economica, incentivando gli investimenti in modo da favorire la riduzione del rapporto debito-PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore. Abbiamo votato, sempre unanimemente, che in questo negoziato si trattasse affinché fossero conciliate le esigenze di una graduale e realistica riduzione del debito. Abbiamo altresì votato che forse - questo era un punto rilevante di quella risoluzione - sarebbe importante andare proprio a rivedere i trattati.

Si è scelto, per la fretta di modificare questo Patto di stabilità e crescita, di non modificare i trattati, che sicuramente è una procedura ben più complessa, ma semplicemente modificare le regole a legislazione data. Il risultato è stato l'approvazione di ieri che ha visto - questa volta sì - l'unanimità di fatto dei rappresentanti italiani, perché PD, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non hanno votato per quella *governance.*

Possiamo parlare di molti dei dati che sono riportati in questo Documento, ma io credo che la politica oggi abbia un imperativo categorico e io sono certa che tutti noi lo sappiamo, visto com'è andato il voto di ieri sul Patto di stabilità. al fatto di rivedere a livello europeo le regole di questa *governance*, perché il tempo dell'austerità lo dobbiamo lasciare alle spalle *(Applausi)* e dobbiamo consentire una crescita delle Nazioni, una crescita di tutti, delle famiglie, di quel ceto medio che il Governo Meloni ha cercato, alle regole date, di sostenere in ogni modo: con il taglio del cuneo fiscale, con la riduzione delle tasse, con i sostegni alla maternità, visto che un altro dei grandi indicatori che ci viene consegnato dall'Istat è impietoso e vede l'Italia, insieme a tutta l'area euro, avere un tasso di natalità bassissimo. Dobbiamo lavorare per incrementarlo, perché le economie che vedono, come la prospettiva ci dice, nel 2050 un giovane a tre anziani non possono crescere. crescere. È anche per questo che ieri mi sono indignata in seno alla Commissione bilancio quando, invece di parlare del PNRR, invece di dissertare su quali potessero essere i moltiplicatori per cercare di rilanciare la nostra economia,

Io credo che forse non ci rendiamo bene conto di quanto sia importante, serio e grave il tempo che stiamo attraversando. Se siamo riusciti ad avere una crescita del tasso di occupazione dei giovani, è stato grazie a sforzi straordinari compiuti da questo Governo, ma è stato anche e soprattutto grazie a qualcosa che contraddistingue e caratterizza l'Italia, cioè la robustezza che è stata dimostrata da quel popolo di piccole e medie imprese, di italiani risparmiatori, capaci di dimostrare sempre elasticità assoluta anche nei momenti duri come quelli che abbiamo dovuto attraversare in questi lunghi mesi e io direi negli ultimi anni. anni. La fiducia è assoluta ed è massima nei riguardi del Governo per il lavoro che continuerà a fare. Spero ardentemente che l'Esecutivo si batterà fino all'ultimo momento nel contesto europeo; sono cosciente che alcune votazioni fondamentali rispetto all'*asset* della *governance* saranno successive alle elezioni europee, che ci vedranno impegnati tutti in questa campagna elettorale e auspico fermamente che possa valere il bene comune italiano, come è accaduto ieri, che ha visto un'unità

un'Europa di lacci, lacciuoli e *austerity*, ma abbiamo bisogno di far crescere nuovamente l'Europa, l'Italia e il nostro popolo.

Freni e mi dispiace che in questo momento non ci sia anche il ministro Giorgetti, perché stiamo parlando del Documento più importante, il DEF, che anticipa quella che sarà la prossima legge di bilancio del Governo. Quello che possiamo evidenziare subito da questo Documento è che non c'è alcuna visione programmatica del Paese, alcuna trasparenza, ma soltanto un Documento che va in direzione contraria rispetto alla fotografia che è stata ben spiegata - lo dicono i numeri, non lo dice il Gruppo di Italia Viva - dai dati Istat nelle scorse settimane: l'inflazione che continua a galoppare, gli stipendi che ovviamente non crescono, mentre crescono e aumentano le tasse. Soprattutto, il dato che ci dovrebbe invece preoccupare tutti, al di là del colore politico, perché parliamo soprattutto di *welfare*, di sanità e di sociale, è che ci sono più di 9 milioni di italiani che si sono indebitati per poter portare avanti le spese mediche necessarie alla cura

Finiamola anche con la retorica dell'aumento delle risorse sulla sanità da parte di questo Governo, perché non c'è nessuna risorsa sull'unica cosa che dovevate fare immediatamente, cioè mettere risorse economiche per assumere nuovo personale medico infermieristico, nuovi operatori sociosanitari, perché quelle risorse in più che avete stanziato vanno soltanto a rinnovare i contratti in vigore del personale esistente e vanno a ripianare i debiti delle Regioni. A questo sono servite quelle risorse in più che ci sono per il Piano sanitario, perché altrimenti ci raccontiamo delle grandi bugie. Allora lo voglio dire qui, perché ne abbiamo parlato anche ieri, con l'intervento di Matteo Renzi e di altri colleghi in sede di esame del decreto sul PNRR, e vale per il DEF e vale purtroppo per tanti altri provvedimenti che affronteremo nelle prossime settimane: vogliamo sì o no invertire la rotta, cercando di stanziare risorse su due priorità, che sono la sanità e l'istruzione? Questi sono due elementi fondamentali per riscrivere le politiche di *welfare*. Oggi non è così. Oggi investiamo il 6,1 per cento del PIL sulla sanità, contro una media europea dell'8 quindi vuol dire che è ancora sottofinanziato il sistema sanitario pubblico. I LEA - lo diceva la collega Lorenzin - non sono stati aggiornati e ancora una volta vi è un rinvio rispetto invece a nuove malattie rare, che non sono coperte dal sistema sanitario pubblico. Questi sono i temi che dovrebbero interessare non solo gli italiani, ma anche il Governo. L'appello

scienziati che chiedono di investire nel sistema sanitario pubblico. Ancora una volta, siccome il Gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe di questo ha fatto una battaglia, la faremo anche in questa campagna per le elezioni europee e anche dopo il 9 giugno, quando avremo i nostri rappresentanti all'interno del nuovo Parlamento europeo. L'Italia dovrà prendere questi 37 miliardi del MES sanitario. Questi sono l'unica cosa importante, che riordinerà

vi sono queste enormi diseguaglianze. Anche tra le Province di una stessa regione e nelle Regioni più avanzate dal punto di vista delle cure sanitarie e dei servizi vi sono dei problemi. Su questo noi abbiamo il dovere di intervenire e su questo non vi sarà mai un approccio ideologico da parte del nostro Gruppo, perché siamo profondamente convinti che serva una riforma del *welfare*. Quando troverete il tempo di parlare realmente dei problemi che riguardano gli italiani, ci troverete al vostro fianco, come abbiamo già fatto in passato. Altrimenti, ci dispiace, ma anche oggi dobbiamo registrare un dato totalmente negativo di un Documento che non è trasparente, che non ha una visione programmatica di quello che accadrà nei prossimi mesi. fotografa il quadro economico esistente e dimostra che, nonostante un momento geopolitico difficoltoso e una crisi energetica perdurante, l'Italia ha dimostrato la sua piena resilienza. È una economia che ha anche reagito al mutare delle condizioni finanziarie, che vedono ancora i tassi della Banca centrale europea alti, per tenere sotto controllo l'inflazione. Lo stanno dimostrando i tassi reali dei prestiti e dei mutui, che, come i rendimenti dei titoli del Tesoro, sono già in calo, anticipando quello che sarà un prossimo taglio dei tassi della BCE. BCE. È un sistema economico che va verso una politica energetica completamente ridisegnata, in direzione dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili, quindi sempre più sostenibile. Eravamo troppo dipendenti dalle fonti fossili e i conflitti nel mondo ci hanno dato una scossa. Il nostro mercato energetico ci ha mostrato come si vada sempre più verso un'economia basata sull'energia *green*, anticipando, in alcuni casi, persino i *target* concordati con l'Unione europea. Gli altri traguardi e obiettivi che si è dato questo Governo sono quelli del PNRR, la cui attuazione sta andando avanti decisa e che darà un contributo importante alla crescita del PIL. È anche aumentata la dotazione complessiva del Piano, che adesso è di 194,4 miliardi; ne rimangono da spendere ben 150 per quest'anno ed i prossimi anni di programmazione. La riprogrammazione degli interventi serve a concludere il piano delle riforme, a superare i molti *gap* del Piano iniziale e a contribuire a un sistema economico più resiliente in molti settori della nostra economia. Anche la pressione sui conti pubblici, a causa della cessione dei crediti dei *bonus* edilizi, ha contribuito a creare un nuovo modello di sostegno pubblico al settore delle costruzioni. Resteranno gli incentivi, ma su livelli sostenibili e mirati a smuovere soprattutto gli investimenti privati, incentivati da un sostegno più pubblico, più logico e calibrato nel tempo. perché l'edilizia, che è un comparto fondamentale, accompagna anche la crescita di molti altri settori. L'Italia sta facendo quello che prima non faceva: revisione della spesa, selezione degli incentivi agli investimenti e delle leve fiscali, un più puntuale utilizzo dei crediti d'imposta. Il Documento di economia e finanza, che non è affatto reticente, disegna questo percorso in oltre 850 pagine, ribadendo i risultati raggiunti a legislazione vigente, e al contempo ci mette di fronte alla possibilità di definire i numeri programmatici sulla base della nuova *governance* europea. Non è poca cosa sapere quale sarà il nuovo piano fiscale strutturale di medio termine, che sostituirà il Patto di stabilità e crescita europeo, e quali saranno i vincoli che ne deriveranno per la nostra economia. nuovo *deficit* del 2023 è stato proprio ieri riclassificato dall'Istat al 7,4 per cento del PIL, soprattutto a causa del superbonus. Intanto prendiamo atto di un'economia che, a causa della pandemia, ha potuto usufruire di una sospensione dei parametri del vecchio Patto di stabilità e crescita europeo. Ma quella gestione a volte disinvolta ora non è più possibile. È necessario continuare con un'amministrazione misurata, che non significa austerità, ma consapevolezza che ogni euro speso vada a buon fine e non venga sprecato. Vanno tenuti sotto controllo gli effetti dei crediti d'imposta, ma ciò non significa privarsi di questo strumento che in molti casi ha avuto un effetto straordinario di stimolo alla crescita. Vorrei ricordare che uno dei sistemi per contrastare l'evasione fiscale è proprio il cosiddetto contrasto di interessi, cioè il cittadino chiede a chi gli fornisce una prestazione la fattura, che ora è anche elettronica (quindi controllabile fin dall'emissione), e l'azienda, ovvero il professionista che fornisce la prestazione, paga la sua parte di tasse. Anche i *bonus* edilizi sono nati con questa *ratio*: lo Stato concedeva il 36 per cento, poi il 42, poi il 50 per cento, di detrazioni fiscali in dieci anni sui lavori per ristrutturare casa e quindi i lavori edilizi facevano emergere un'economia e soprattutto tutelavano i lavoratori, perché lavoravano totalmente in regola. L'anomalia è stata innanzitutto quella di mettere in campo percentuali troppo generose di detrazioni, come il superbonus 110, in questo modo perdendo il moltiplicatore del contributo pubblico all'investimento privato, che deve appunto partire dal cittadino privato contribuente. Poi fa perdere il controllo sul valore reale dell'investimento: in molti casi, anche dove non ci sono state truffe evidenti, si è arrivati a un valore di lavori del 110 per cento molto più alto rispetto al vero valore dei lavori reali. Altro errore è stato quello di consentire lo sconto in fattura, posto che pochissime imprese edilizie hanno una tale capienza fiscale per tutto l'anno da poter assorbire i crediti, e soprattutto la cessione multipla del credito, che ha fatto perdere completamente il controllo della situazione. Il credito d'imposta deve tornare ad essere una leva fiscale per incentivare gli investimenti privati e per far emergere il nero. Nel settore dell'edilizia è fondamentale evitare quel sommerso che inevitabilmente genera anche lavoro nero, quindi minore sicurezza per i lavoratori. Il Documento espone comunque un quadro a legislazione vigente con dati di tutto riguardo (specie rispetto agli altri Paesi europei), che presuppone numeri buoni sulla tenuta della nostra economia, una volta che verrà ultimata la programmazione per il triennio. Per questa ragione apprezziamo il lavoro finora svolto dal ministro Giorgetti; lavoro che verrà traslato nelle nuove regole europee del piano fiscale e strutturale di medio termine con basi solide. C'è la consapevolezza di avere numeri sotto controllo per proseguire sul solco già tracciato dalla legge di bilancio dello scorso dicembre, all'insegna del sostegno alle famiglie e ai lavoratori, della facilitazione a investire e a creare posti di lavoro, cioè fare quello che deve fare uno Stato: dettare regole chiare, semplificare l'iniziativa privata, anche incentivandola per raggiungere l'obiettivo di far crescere l'economia.

oggi non siamo chiamati a votare veramente sul DEF, ma a partecipare a un importante esercizio di sospensione, trattenendo il fiato, devo dire. Sospensione dovuta in parte ad alcuni elementi di incertezza del quadro istituzionale e politico europeo, che sono stati giustamente sottolineati. Ma la parte più insidiosa del clima di sospensione è - ahimè - *made in Italy*, fatta in casa, e ha due componenti: una componente generata nel passato e una componente che, temo, stiamo generando in questi mesi e in questi giorni, convinti di servire l'interesse del nostro Paese. La componente generata nel passato è naturalmente il debito pubblico. Io non vedo sufficiente consapevolezza del problema del debito, né sufficiente volontà di affrontarlo, come temo, anzi sono certo, prima o poi sarà duramente necessario. Questo è un rilievo che muovo sì al Governo, ma forse ancora di più alle opposizioni, che, se andassimo a calcolare i millesimi di responsabilità nella generazione per esempio del superbonus (sarebbe un esercizio facile e utile anche pedagogicamente), con i due Governi precedenti a quello attuale, ai quali non partecipava il partito di maggioranza relativa dell'attuale maggioranza, hanno fatto ben al di là di quello che si pensava umanamente fattibile in termini di generazione del disavanzo. Hanno fatto qualcosa di molto ardito anche sul piano equilibristico, perché in un Paese nel quale, come è noto (giusto o sbagliato), è mortale pronunciare la parola "imposta patrimoniale", tutti coloro che hanno votato per il superbonus hanno votato (spero per loro senza saperlo) per un'imposta patrimoniale sulla casa però al rovescio, cioè con il contribuente che paga un trasferimento di ricchezza ai proprietari di casa, i quali mediamente hanno una situazione di reddito e di ricchezza migliore di quella del contribuente. Questo ha determinato una grossa redistribuzione perversa del reddito, proprio sotto ogni profilo che si possa immaginare. Leggevo ieri un articolo che spiegava come, oltre alle conseguenze sulla finanza pubblica e oltre alle conseguenze di questa imposta patrimoniale al rovescio, si è statisticamente appurato che i benefici maggiori del superbonus sono andati alle rendite e al Nord, proprio come uno si aspetterebbe da un provvedimento nato con questa lungimirante concezione di giustizia sociale. La seconda componente del disagio che io avverto, e che sinceramente spero ogni collega avverta e ogni Gruppo parlamentare senza eccezione avverta, perché credo che comincino ad avvertirla i nostri concittadini e che comincino a vergognarsene, condotta complessiva del nostro sistema Italia, di cui siamo giustamente orgogliosi (e qui ce lo diciamo, moltiplicando a vicenda il nostro orgoglio di essere italiani): stiamo mostrando una disconnessione pazzesca fra le componenti del sistema Italia agli occhi dell'Europa. Come è stato già accennato, siamo l'unico Paese i cui eurodeputati, di maggioranza e di opposizione, si siano si siano astenuti in blocco o abbiano votato contro le regole di bilancio. Non ho scrupoli. So che molti di voi amano, magari come una forma di cilicio espiatorio, l'austerità, mentre a me non è mai piaciuta, tant'è vero che, intervenendo in Senato a dicembre, avevo suggerito alla Presidente del Consiglio, in vista di quel Consiglio europeo finale di dicembre, di considerare seriamente se non fosse il caso, da parte dell'Italia, di porre il veto a quell'accordo poco soddisfacente sulla nuova *governance.* È stato deciso di non porre il veto e adesso, se voi foste un cittadino di un altro Paese europeo che ama l'Italia come noi, che impressione avreste? Qualche mese fa,

e che occorre il processo di ratifica, si è rifiutato di avviare tale processo anche se gli sono stati porti su un vassoio strumenti di minimizzazione del rischio (tipo, si chieda la ratifica con la condizione che il Parlamento debba di nuovo pronunciarsi ove mai il Governo intendesse fare uso di quegli strumenti). Pertanto, siamo disconnessi sul piano del MES. signore e signori, siamo disconnessi sul piano del più importante strumento di *governance* europeo, al quale muovo molte critiche e avevo suggerito al Presidente del Consiglio di opporsi. Ma adesso cosa succederà? Quando il Presidente del Consiglio, che ha affermato, rispetto al punto di partenza, una - credo - forte complessivamente buona e coerente immagine in Europa, andrà alla seduta del Consiglio europeo che dovrà chiudere in bellezza questo pacchetto (che a me non piace) che cosa dirà o farà, aderendo, perché richiede l'unanimità, alla posizione di tutti i suoi colleghi, un torto agli europarlamentari del suo Paese, o alimenterà, ancora, una plateale immagine di inaffidabilità del nostro Paese? Io vorrei che, anziché votare (per carità, dobbiamo farlo; io non lo farò, ma sono in una posizione fortunatamente particolare) un DEF che non è un DEF, ragionassimo un pochino di più su questa situazione in cui siamo messi e ci stiamo mettendo. Concludo, Presidente, dicendo che quando il Governo italiano, italiano, il Parlamento italiano, autorevolissimi - e più d'uno - *ex* Presidenti del Consiglio italiano che scrivono rapporti per le autorità europee, parlano positivamente della necessità di creare un debito europeo, ma chi volete che creda a loro, al di là della loro autorevolezza personale? Da quale Paese vengono? Vengono dal Paese che noi rappresentiamo qui e nell'altra Camera e che è guidato da Palazzo Chigi. Cerchiamo di riflettere se l'Europa sia perversa, prevenuta contro gli italiani, o se noi non stiamo assumendo anche adesso che abbiamo capito quanto importante sia l'Europa - dei comportamenti sciatti, controproduttivi e tutto sommato indegni.

colleghe e colleghi, è inutile che ricordi a tutti noi quanto sia importante la sanità, anche se i più se ne ricordano solo quando qualche evento avverso tocca da vicino. Io me ne occupo quotidianamente e se dovessi dire di essere soddisfatta di cosa e di quanto prevede il Documento di economia e finanza dovrei essere menzognera. Ma vero è che dobbiamo essere pragmatici e il realismo ha sostanzialmente imposto di agire per far sì che venga a essere suonata la campanella della fine ricreazione a fronte del debito monstre tendente ai 3.000 miliardi. Fortunatamente abbiamo un Governo responsabile e non c'è bisogno che gli venga ricordato che bisogna rientrare nei parametri.

che paiono immutabili, ma diciamo pure che gli anni difficili della pandemia sono una giustificazione almeno parziale. Con la pandemia, c'è stato anche un periodo di crisi energetica tale per cui alcuni costi sono andati fuori controllo sia per le aziende pubbliche e private, che per i fornitori di beni e servizi. Superato il momento di picco e fermi ulteriori scenari di guerre, per reperire nuove risorse in sanità - e Dio solo sa quanto ce n'è bisogno - dovremmo cercare prima di individuare dove è possibile razionalizzare, perché per esempio, se è vero che da una parte vi sono nuove e più performanti soluzioni terapeutiche che inevitabilmente pongono un problema di risorse, altrettanto vero è che, dall'altra, dobbiamo tener conto di tutti quegli sprechi che ancora si annidano nei meandri del sistema, per esempio andando a verificare in tempo reale se le prestazioni richieste sono ancora nell'interesse di chi a suo tempo le ha prenotate, dato che quasi il 25 per cento non si presenta agli appuntamenti e questo è uno spreco che non porta vantaggio a nessuno e in caso contrario, scorrere le graduatorie. Altrettanto vero è che il nostro servizio sanitario è apparentemente uno dei meno costosi se paragonato in termini percentuali rispetto al PIL di altri Paesi a noi assimilabili, ma ancor più vero è che vi è una spesa *out of pocket* di cui non abbiamo piena contezza, a cui dovremmo sommare 11 miliardi di costo che

Io sono certa che il nostro Servizio sanitario nazionale sia uno dei migliori in senso assoluto, specie per la vocazione universalistica che gli è propria, ma che, come tutte le cose, anche le migliori, necessiti di qualche revisione dovuta alla storicizzazione di alcuni problemi e al ritardo nell'evoluzione della capacità di risposta ai nuovi bisogni. È per questo che mi sono permessa di richiamare più volte anche alla vostra attenzione l'importanza di intervenire con nuove direttrici di natura sia ordinamentale che settoriale, a cominciare dalla riorganizzazione dell'emergenza urgenza pre-ospedaliera ed ospedaliera, che, in combinato disposto con il riordino della medicina territoriale, andrebbe a disintasare i pronti soccorso degli ospedali, implementando modelli innovativi di presa in carico dei pazienti, secondo percorsi preventivo-diagnostico-terapeutici mirati e personalizzati. Il contrasto delle inappropriatezze prescrittive, infatti, non può essere disgiunto dall'agire in prevenzione. Per questo sostengo che la prevenzione predittiva e proattiva sia il futuro della nostra sanità. Non è solo una mia affermazione, ma recenti studi ci ricordano che ogni euro investito in prevenzione genera quasi quattro euro di valore in termini di benefici individuali e collettivi. Uno dei punti su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è un altro investimento in prevenzione ed educazione sanitaria di lungo periodo, che ritengo molto importante, vale a dire che nelle scuole primarie e secondarie si abbia un medico di istituto che vada a individuare precocemente i problemi degli alunni; reclutabile con strumenti selettivi, innovativi e attrattivi per i giovani medici. Mi rendo conto

di investire in un patto generazionale con docenti e famiglie, per avere nuove generazioni consapevoli di quanto sia importante la prevenzione. Loro stessi, che abbiano ad aver avuto prova della sua centralità, saranno degli adulti sani e degli anziani non solo longevi, ma in buona salute, con conseguenti risparmi in cura. Conclusivamente ne discende che dovremmo immaginare di utilizzare risorse di altri capitoli di spesa nella prossima manovra di bilancio, da finalizzare per le priorità di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva, con meccanismi di valutazione e di controllo di tracciabilità degli impieghi e degli esiti, che ci vedano tutti trasversalmente impegnati in innovazione e cambiamento.

c'è il Patto di stabilità. L'unico Gruppo a votare contro il Patto di stabilità è stato il Movimento 5 Stelle. Eppure voi prima gridavate che la pacchia era finita in Europa: una volta che noi andremo al Governo, la pacchia sarà finita. Invece adesso avete supinamente accettato il Patto di stabilità.

colleghi, io potevo anche accettarle se in campagna elettorale aveste detto qualcosa di diverso. Invece voi avete detto tutto e il contrario di tutto e oggi quelle misure che avete difeso urlavate contro l'Europa - sono completamente svanite.

a febbraio 2021, pesava zero. La nostra legge, per come l'abbiamo scritta noi, nel dicembre 2021 pesava 16 miliardi da distribuire in cinque anni:

sul superbonus, oltre 200 modifiche sui bonus edilizi da quando l'avete gestito voi. Allora, quello non è più il nostro superbonus, quello è il vostro superbonus. E non vi abbiamo mai sentito dire dovesse essere modificato in modo strutturale, abbassando quella percentuale che era da pandemia del 110 per cento. Noi avevamo previsto un *décalage*, ma non l'abbiamo potuto fare perché non eravamo più al Governo.

2021, in cui pesava 16 miliardi, siamo arrivati al Governo Meloni che pesava 50 miliardi. Da quando siete insieme, inclusi Fratelli d'Italia, è arrivato da 50 miliardi a 120 miliardi: 70 miliardi sono vostri, li avete causati voi, li ha causati il ministro Giorgetti *(Applausi)*. Di quei 70 miliardi che sono andati soprattutto nelle tasche degli imprenditori padani, che oggi chiamate ladri e furbi, 22 miliardi sono andati in Lombardia,

Com'è che avete 18 miliardi per un ponte inutile? Sapete che gliene frega del Ponte sullo Stretto all'imprenditore veneto? Nulla. Ecco perché non esistete più, state scomparendo. E chi vi sta rubando i voti? Il vostro compagno di coalizione che dice di essere a favore del superbonus, ma Giorgetti glielo nega. Voi avete questi due Ministri che sono i gemelli dell'autogol, Giorgetti e Salvini, che vi stanno distruggendo,

sono uno di quelli vicini alle imprese, sono uno di quelli del MoVimento che parla con le imprese venete e lombarde e vi assicuro che l'imprenditore padano la Lega non la può più vedere per questo, perché state dando i soldi al Ponte sullo Stretto, di cui non frega niente a nessuno, e avete tolto i soldi che hanno arricchito il Nord, hanno capitalizzato le banche del Nord. Bravi, bravissimi, un'operazione vincente.

Salvini e Giorgetti, vi stanno facendo sparire e i sondaggi lo dicono. *(Commenti)*.

Se vi fosse stato un cosiddetto *décalage*, così com'era previsto dalla misura ideata dal MoVimento 5 Stelle, le imprese avrebbero investito nelle catene produttive, avrebbero visto una pianificazione a dieci o quindici anni ed il PIL sarebbe cresciuto ancora di più.

in Italia, col superbonus, è cresciuto di soli tre punti. Quindi, dove non c'è stato il superbonus, in Paesi post pandemici come noi, il debito è aumentato. Perché in Italia, col superbonus, il debito è cresciuto meno degli altri Paesi? Evidentemente perché il superbonus ha generato un effetto positivo sul PIL e quindi il rapporto debito PIL ne ha tratto un beneficio. Per questo, voi capite che tutto quello che avete detto, grazie ai media che ormai sono tutti nelle vostre mani, dai giornali alle televisioni, e parlano male di questa misura, sono solo bugie e gli imprenditori lo sanno. Voi potete prendere in giro qualche sprovveduto, ma il sistema produttivo italiano vi ha capito. Quando parlo con gli imprenditori, questi sanno benissimo che il disastro l'ha combinato Giorgetti. Egli gestisce questa misura dal febbraio 2021 ad oggi: oltre tre anni e mezzo di superbonus gestito dalla Lega. Tutto quello che è successo è solo colpa vostra. Avevate una misura così ampia e forte da farci uscire dalla crisi pandemica, che dovevate semplicemente rendere

Governo ad oggi, i 70 miliardi in più di peso del superbonus in più generati da voi, dal vostro panico, dalle vostre paure, dalle vostre bugie non ci sarebbero stati. Fatevi, dunque, un esame di coscienza. State portando il Paese alla deriva. State distruggendo la nostra economia e non ve ne state rendendo conto.

cento del superbonus è relativo al Governo Meloni. Il Governo Conte II è finito a gennaio 2021.

onorevoli senatori, iniziamo subito a sgomberare il campo dalla critica più infondata che ho sentito nelle ultime settimane, e cioè che un Documento di finanza pubblica secondo molti ridotto all'osso non sarebbe degno di essere valutato in questo Parlamento. all'esito di un negoziato complesso - non a caso non abbiamo votato - sulla proposta della Commissione europea in seno al Consiglio Ecofin, è stata convenuta una vera e propria riforma a livello di trilogo, il Parlamento europeo ieri ha approvato definitivamente le nuove regole. Quindi, il primo passo della nuova *governance* del Patto consisterà nell'invio entro il 21 giugno, da parte della Commissione, di un percorso di riferimento per definire un profilo temporale di crescita massima dell'aggregato di spesa pubblica netta, in base al quale gli Stati membri dovranno costruire i *medium-term fiscal structural plans*, ossia i futuri piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine. Perciò la scelta del Governo di presentare un DEF tendenziale denota, oltre che rispetto - ahimè - degli impegni presi con l'Europa, anche serietà e pragmatismo. Poiché troppe volte ho visto scarsissima memoria su questo, mi preme anche ricordare che non è la prima volta che il DEF ha solo le stime tendenziali: ci sono stati già ben quattro precedenti e anche in ambito europeo l'Italia non sarà l'unico Paese a presentare un Documento di finanza pubblica semplificato, proprio per la natura di transizione delle nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025. Per chi invece avesse perso anche la vista, riguardo a ciò che concerne il *deficit*, oltre al netto dell'impatto sui conti pubblici del 2023, causato dall'ulteriore aumento dei costi legati al superbonus, le tendenze delle principali grandezze sono in linea con quelle previste dallo scorso settembre nella NADEF. Il nuovo sistema di regole è maggiormente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica, e in particolare della spesa primaria e del relativo monitoraggio. Una valutazione attenta dell'entità dello sforzo fiscale che sarà richiesto con l'entrata in vigore del nuovo sistema ha portato il Governo a dare conto, in questo Documento, del fatto che gli andamenti programmatici futuri non potranno che essere individuati al più tardi entro il 20 settembre di quest'anno. Entro il 20 settembre perciò l'Italia dovrà presentare - e presenterà, state tranquilli - il nuovo piano strutturale di bilancio di medio termine, con un orizzonte quinquennale e un particolare riferimento all'andamento della spesa primaria netta. Alla luce di queste considerazioni, è evidente che non era necessario definire nel DEF degli obiettivi diversi dalle grandezze di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale a legislazione vigente, e che allo stesso tempo si è riportata una stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà priorità rifinanziare il taglio del cuneo fiscale sul lavoro. Inoltre, questa maggioranza ha la volontà di continuare ad intervenire sul profilo del *deficit*, migliorandolo ulteriormente anche attraverso una revisione della disciplina dei crediti d'imposta, al fine di ricondurlo al di sotto del 3 per centro entro il 2026 e a non discostarsi dai valori della NADEF anche per gli anni 2025 e 2026. Un forte impulso della crescita del PIL sarà sostenuto dal tanto criticato - lo abbiamo visto anche ieri - PNRR e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie, tenuto conto che l'azione del Governo per il 2024 è proseguita proprio in tale direzione. Il sostegno ai redditi dei lavoratori, avvenuto prevalentemente tramite la riduzione contributiva, ha consentito anche di moderare la spinta salariale, volta al recupero del potere di acquisto. Concludo. Le numerose critiche che abbiamo sinora ascoltato, in realtà - lo sapete benissimo anche voi, ma lo sottolineiamo e lo ricordiamo - vanno addebitate alle scelte dei Governi precedenti, compreso il superbonus, questo sì con il rischio di farci piangere per tutta la prossima generazione. Finalmente c'è un Governo che basa la sua azione non sui soli sussidi, ma sulla crescita e sullo sviluppo. È finito il tempo dei numeri dati a caso, come proprio per il superbonus; così come è finito il tempo della gestione allegra delle casse pubbliche. Al modello passato della sinistra, fatto di sussidi a pioggia e redditi di cittadinanza, il Governo Meloni ha finalmente contrapposto il modello della responsabilità e dell'equità. È così che questa maggioranza affronta una fase difficilissima: investendo su famiglie, lavoratori e imprese. Grazie alle nostre misure, con la maggioranza di centrodestra siamo credibili e rispettati anche in Europa. Il Governo Meloni è stato capace di tenere alti lo *standing* internazionale e la capacità di crescita della Nazione. Il prossimo G7 giugno ne darà un'ulteriore dimostrazione.

Presidente, saluto il sottosegretario Freni. Cari colleghi, se si parla di conti pubblici, come non si può cominciare con l'angoscia causata dal disastro del superbonus? Come non rimarcare, proprio qui, le parole del ministro Giorgetti, quando ha detto che il superbonus si è mangiato un anno intero di incrementi della spesa sanitaria? Come non pensare poi che questa tragedia contabile graverà in maniera inesorabile sulle spalle degli italiani per i prossimi anni, se non addirittura per i prossimi decenni? Giustamente sempre il ministro Giorgetti, intervenuto in Commissione bilancio, ha ricordato come il Governo ha dovuto tenere conto delle possibili ripercussioni del complesso contesto geopolitico internazionale, improntando le previsioni a un principio di cautela e di prudenza, Si sono dovuti tenere in conto le guerre in corso, le tensioni in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina, l'instabilità delle rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e quant'altro. Proprio considerando il quadro geopolitico in continuo mutamento e a seguito di un corretto ragionamento sulla strategicità degli investimenti in difesa, con il raggiungimento del 2 per cento del PIL per la difesa nostra e dei nostri alleati,

al totale della spesa dei bilanci per la difesa - ma, attenzione - non del nostro Paese però, non dell'Italia. È equivalente ai bilanci della spesa per la difesa di tutti i Paesi europei messi assieme. Non solo. Sempre per fare un paragone, il Fondo sanitario nazionale finanziato dallo Stato quest'anno vale 36 miliardi, contro - non mi stancherò mai di ripeterlo - gli oltre 220 miliardi del superbonus. Senza poi contare le migliaia di truffe e di irregolarità accertate ormai inequivocabilmente dall'Agenzia delle entrate. Bene, mi verrebbe da dire, ma invece è male. Giusto per farci un'idea più chiara di cosa abbiamo davanti, in in questo contesto particolarmente complicato, articolato e difficile, il DEF e le politiche del Governo cercano, nonostante tutto, di essere realiste, pragmatiche e concrete. Concordo anche sul fatto che il consolidamento della finanza pubblica rappresenta davvero una sfida, che dovremo affrontare assieme al Governo e al Parlamento in maniera assolutamente strategica e sinergica. La sfida è grande, ma riteniamo che l'aggiustamento sia assolutamente alla nostra portata. Ricordo infine come, a proposito proprio di conti pubblici,

cui la Lega è protagonista attraverso i suoi Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari, ad aver denunciato la follia del superbonus, mettendo la parola fine a questo enorme spreco. Questo, insieme alle politiche portate avanti, ci fa avere fiducia nell'Esecutivo e nella stagione della nostra economia, con l'auspicio che anche le situazioni contingenti negative possano finalmente terminare, dando ossigeno alla nostra economia, al nostro Paese e, soprattutto, alle tasche degli italiani, che tanto e troppo hanno sofferto a causa della grave crisi. *(Applausi)*.

io ritengo che la discussione che stiamo svolgendo oggi in Aula sia fortemente destituita di dignità dalla scelta operata dal Governo di presentare al Parlamento - e al Paese, di conseguenza - un DEF sostanzialmente politicamente muto rispetto agli impegni programmatici che un Esecutivo, nel pieno delle sue funzioni e a metà del suo mandato, dovrebbe indicare.

avrebbe il dovere di indicare al Paese e al Parlamento quali sono gli indirizzi di politica economica e fiscale e gli interventi di politica industriale per la crescita che intende portare avanti. avanti. Presidente, non ne faccio una questione formale di ottemperanza o meno alla legislazione vigente sulla finanza pubblica, tema che pure è stato sollevato da diversi colleghi anche lunedì sera, durante l'audizione del ministro Giorgetti a Montecitorio. faccio una questione propriamente e squisitamente politica, perché crediamo che il compito e il dovere di un Governo sostenuto da una maggioranza solida siano quelli di tracciare una via non soltanto nella discussione parlamentare,

all'economia e agli investitori internazionali per indicare quali sono la strada e la strategia che il Paese intende adottare da qui ai prossimi mesi. Nulla di tutto ciò è possibile valutare in questo Documento che - come è noto - si limita a prendere atto dell'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e a indicare un quadro tendenziale, a legislazione vigente, per gli esercizi futuri. Quello che sappiamo, invece, ci preoccupa. Possiamo giudicare e valutare come le stime di crescita che il Governo ha indicato nel Documento siano poi state corrette al ribasso - ahimè dai grandi osservatori e dalle autorità indipendenti, come Banca d'Italia ed Eurostat. A fronte di stime che il DEF individua tra l'1 e l'1,2 per cento per gli anni futuri, Banca d'Italia ed Eurostat prevedono una crescita che oscilla in una forchetta ben più ridotta, compresa tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento. Altra cosa rilevante e che non possiamo che giudicare con preoccupazione è il fatto che, in assenza degli investimenti dovuti al PNRR, la nostra economia sarebbe in stagnazione, se non addirittura in recessione, come indicato dai dati tendenziali del Documento. L'unico apporto alla crescita è quello del PNRR, su cui abbiamo discusso ieri. Troviamo l'azione del Governo non incisiva, né convincente nello spingere questo importante Piano. D'altra questa considerazione porta a evidenziare come le politiche per la crescita attuate nei diciotto mesi di Governo siano state del tutto insufficienti a generare qualche impatto significativo sulla traiettoria del nostro PIL. E sono state insufficienti perché non non ve ne sono state. Non abbiamo discusso in quest'Aula di alcun provvedimento che parlasse di investimenti, di politica industriale, di strategia a sostegno di campioni nazionali, delle grandi, delle medie e delle piccole imprese del nostro territorio.

come è noto - questo è previsto in crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali, tra cui ovviamente quelli per l'efficientamento energetico. L'andamento della spesa per il superbonus, che è indicato nel DEF come principale responsabile dell'aumento del debito, è in realtà un aumento di costi che è spalmato su ben quattro anni di vigenza di questo provvedimento; quattro anni dei quali quasi due sono stati gestiti dal Governo guidato da Giorgia Meloni e dal ministro dell'economia Giorgetti *(Applausi).* E quindi non può valere a giustificazione del Governo, che ha avuto tutto il tempo di provvedere con appositi provvedimenti, che pure abbiamo discusso e votato, ad aggiustare il tiro rispetto ad un provvedimento che ha visto sicuramente degli elementi positivi, anche di impatto sulla crescita del Paese, ma che andava - come diremo nella discussione delle prossime settimane - rivisto e riportato in una traiettoria in grado di essere compatibile con i parametri della finanza pubblica.

è dove troverà il Governo quei 20 miliardi necessari a sostenere le misure che abbiamo approvato in una legge di bilancio composta in gran parte da misure finanziate per un anno solo, a partire dalla delega fiscale. Non si è mai vista, in questo Paese, una riforma fiscale che valesse per un solo anno e che avesse una copertura di un solo anno. Ma sono diverse le misure che hanno una copertura così ristretta, a partire da quella assai rilevante per i cittadini e e di indubbia rilevanza politica che è la riduzione dell'abbattimento del cuneo fiscale. Nulla ci dice in proposito questo Documento e quindi oggi votiamo senza sapere come il Governo coprirà i circa 20 miliardi. Quello che si capisce, invece, dalle stime tendenziali è una volontà di andare ad incidere sulla spesa, sulla spesa, che significa riduzione degli investimenti nella sanità e nella previdenza e questo elemento ci preoccupa in particolar modo. Il DEF indica questa direzione nei servizi per i cittadini, che non soltanto significa una mancata offerta di accompagnamento e di sostegno soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, ma che per contribuire ad erodere il potere d'acquisto dei cittadini. Quando un servizio come la sanità non viene offerto dallo Stato, significa che per curarsi è necessario rivolgersi alla sanità privata e non bastano 80 euro *una tantum* di mancetta nella tredicesima per compensare compensare la spesa che si deve sostenere per una sanità dignitosa. *(Applausi)*. Veniamo così al nodo più rilevante, almeno per quello di cui mi occupo in Commissione finanze con tanti colleghi, ovvero l'attuazione della delega fiscale. Il Governo ha fatto della battaglia fiscale una bandiera di ordine politico. Ho detto che non è chiaro come verrà sostenuta e finanziata la riduzione delle aliquote fiscali. Siamo in attesa di leggere il nuovo testo che ha tutto il sapore di un provvedimento *last minute* che precede le elezioni, la campagna elettorale. Sui parlato di un provvedimento ancora una volta *una tantum* - promesso per tutti ma in realtà destinato a pochi - di aumento della tredicesima per circa 80 euro. Tutte queste misure frammentate, estemporanee e finanziate a singhiozzo non non vanno però ad incidere sui veri problemi del nostro sistema fiscale; problemi che hanno a che fare con un dualismo esasperato tra chi paga l'IRPEF e chi accede a regimi separati e regimi cedolari, essendo in realtà documentato dai dati che chi paga l'IRPEF è una minoranza di contribuenti che sostiene la maggioranza delle entrate fiscali del Paese. Dopo tutta questa propaganda, questa indicazione di rotta sbagliata sui temi fiscali, sapete, colleghi e colleghe, qual è la notizia che il DEF ci consegna? Tutti questi provvedimenti, annunciati come modalità di introdurre un fisco amico e di ridurre la pressione fiscale, in realtà - come denuncia il Documento che oggi ci apprestiamo a votare non fanno altro che aumentare la pressione fiscale. Il DEF ci dice che nei prossimi anni la pressione fiscale aumenterà dello 0,3 per cento. Quindi domando a me stessa e ai colleghi esattamente che idea di Paese, che idea di patto fiscale che sostenga un patto sociale ci sta proponendo questo Governo. È un'idea un po' furbetta, un po' furbesca che promette tagli e riduzioni o sconti anche di sanzioni,

il Documento di economia e finanza è uno dei tre strumenti di finanza pubblica sui quali si fonda la politica economica del Paese; è uno dei tre strumenti fondamentali, è quello che ci dice cosa vuole fare il Governo.

era già qui, era già seduto e si era alzato; per carità, nessuno vuole impedire al Sottosegretario di spostarsi e poter parlare, ma è indubbio che il Documento di economia e finanza sia un atto così importante che avrebbe richiesto la presenza del Ministro. Non me ne voglia il sottosegretario Freni, non è una questione personale, ma credo che mai come in questa occasione e davanti a un DEF come quello che ci è stato presentato sarebbe stato necessario che il ministro Giorgetti ci mettesse quantomeno la faccia e venisse a a discutere in Aula col Parlamento, cosa che purtroppo evidentemente ha scelto di non fare. Dico questo perché quello che è stato presentato - come abbiamo detto più volte e nel dibattito d'Aula è già emerso e rischio di ripetermi - - è un DEF tendenziale, non è accompagnato da un quadro programmatico, non ha un'indicazione di cifre, cioè è un atto quasi di fiducia, come lo ha prima definito anche il senatore Monti. Si tratta di una sospensione delle nostre attività che ci chiama a fare una manifestazione di fiducia, perché, non essendoci cifre, dobbiamo limitarci ad accettare o meno quello che ci viene narrato, raccontato. Questo è grave, perché chiaramente il Parlamento si esprime sulla base dei numeri e di dati oggettivi che servono a valutare la fondatezza dell'idea che il Governo dà della propria programmazione economica. L'assenza dei numeri ci impedisce di fare questa valutazione in maniera compiuta, di avere un riscontro oggettivo di ciò che siamo chiamati a fare.

di sostegno all'economia e poi non indicare dove si troveranno le risorse per sostenere tali misure. Mi riferisco chiaramente al cuneo fiscale; già nella precedente legge di bilancio era stata prevista l'introduzione del cuneo fiscale per un anno. per un anno. Già questo ci aveva allarmato, perché non si può pensare di ridurre il cuneo fiscale con una misura che ha una durata temporanea di un anno, perché non ha impatto dal punto di vista strutturale, anzi determina anche da parte dei contribuenti un'incertezza su quelle che saranno le loro risorse. Adesso ci viene promesso che sarà rinnovata per un altro anno, così come le aliquote Irpef, che sono state ridotte con la precedente legge di bilancio e con quella vigente. Ci viene detto che anche questa misura sarà rinnovata per un altro anno, ma queste non sono misure che che hanno un impatto strutturale, sono sempre temporanee. L'assenza di una politica strutturale, dal punto di vista economico e finanziario, si traduce nei fatti in mancanza di fiducia da parte dei consumatori, da parte dei cittadini. Lo vediamo nella realtà, è inutile che stiamo qui a fare teoremi di finanza pubblica pensando di essere più bravi degli altri. La realtà dei fatti la vediamo nel carrello della spesa, perché quando i prezzi continuano ad aumentare, invariato il salario e aumentano anche le imposte indirette, che questo Governo ha aumentato, la conclusione è chiara: il cittadino si è impoverito. Qualsiasi stima, qualsiasi proiezione che viene fornita da questo Governo viene smentita dagli indici Istat: il carrello della spesa cresce, il salario rimane invariato. Ciò vuol dire che il costo della vita è aumentato e, a fronte di un costo della vita che aumenta, il Governo non ha risorse, non mette in piedi nessuna politica di programmazione strutturale *(Applausi)*, non incide sul *trend* deficitario crescente. DEF al nostro esame che cosa ci dice? Quali sono le risorse sulle quali il Governo punta per spingere l'economia per questo rilancio? Nessuna, se non il PNRR; questo PNRR è una sorta di coperta, infatti serve a coprire un po' tutto per questo Governo, tant'è vero che già si sa ed è allo studio la proroga delle scadenze del PNRR, perché, con la motivazione che non si riuscirà probabilmente a rispettare queste scadenze al 2026, si dice: non perdiamo l'occasione, non perdiamo le risorse del PNRR, proroghiamo le scadenze al 2028. Astrattamente, è un discorso anche sostenibile, ma nella sostanza tradisce una sostanziale incapacità da parte del Governo a reperire le risorse, sicché questa coperta cerchiamo di stirarla quanto più possibile e farla arrivare fino al 2028. Peccato, però, che più si allungano le scadenze del PNRR, più ovviamente il rapporto tra la risorsa PNRR e il PIL e il PIL varia in senso negativo, perché, se invariate sono le risorse, ma devono durare più a lungo, chiaramente si vanno riducendo anno per anno. Allora, un DEF che non tiene conto di questo, che non ci dà risposte, che pensa di buttare sempre la questione sul superbonus, attaccandolo come se fosse l'unico male dell'economia nazionale, è veramente è veramente miope. Tra le cose sulle quali ritengo che si debba veramente accendere i fari e chiedere al Governo di essere preciso e dare dati certi, vi è la raccolta straordinaria fatta con gli strumenti della rottamazione. La rottamazione è uno strumento che è stato accolto con grande favore dagli elettori e ben venga, anche perché il tasso degli interessi e delle sanzioni economiche in Italia è altissimo e davvero rende l'imposizione quasi insostenibile; questa è la motivazione per la quale c'è una evasione storica

pagherà le tasse dell'anno corrente. Tutto, infatti, sarà rinviato ad un momento successivo, quando ci sarà una rottamazione, questo mio debito verso lo Stato verrà ridotto e io potrò accedere ad altri benefici

è il momento di pensare realmente a una riforma tributaria, a una riforma del sistema dei tributi, che certamente non può essere affrontata con una riduzione delle aliquote Irpef rinviata da un anno all'altro. Quindi, questo DEF è uno strumento che non non risponde veramente alle sue finalità. La discussione odierna non consente al Parlamento di esprimersi chiaramente. L'abbiamo detto già in occasione della discussione della legge di bilancio: la manovra presentata a dicembre del 2023 è carente. Serve una media di 18 miliardi di euro di risorse da reperire per sostenere effettivamente la manovra di bilancio. Dove le reperirà il Governo? Quando le reperirà? Evidentemente dopo il DEF e dopo le elezioni europee.

signori del Governo, colleghi, io vorrei avere dei giudizi meno caustici sul Documento di economia e finanza, ma mi pare evidente, dai numeri e dalla snellezza del provvedimento, che la maggioranza si sta solo nascondendo dietro questi pochi dati in vista delle prossime elezioni europee, per non ammettere che alle promesse fatte agli elettori mancano "solo" venti miliardi o poco meno: quelli che servirebbero per confermare il cuneo fiscale, la revisione delle aliquote Irpef e qualche altra promessa fatta qui e là nel corso degli ultimi mesi. questo è quello che non c'è scritto, ma che, ad uno sguardo attento, emerge chiaramente, come hanno evidenziato già anche altri colleghi prima di me. Cosa ricaviamo da questo Documento di economia e finanza? Che non avete una visione per il Paese e, se la avete, non è certo positiva per i cittadini italiani. Dalle audizioni che sono state fatte nei giorni scorsi è emerso chiaramente che abbiamo tanti problemi. Il primo, di natura economica, è che c'è di nuovo una contrazione del credito alle imprese, lamentato da più parti. Le banche fanno extra profitti, li tengono caldamente in pancia e non erogano fondi all'economia reale; salvo, poi, alzare gli interessi sui depositi nei conti correnti dei deputati alla Camera, forse per ringraziare delle modifiche alla norma sugli extraprofitti. Chissà: a pensar male si fa peccato, ma... Quindi, l'economia reale non la sosteniamo, di sicuro non con il credito. Abbiamo chiesto al Ministro cosa pensasse di fare per aiutare, ma la risposta non è pervenuta, quantomeno in audizione. Chissà se oggi il Governo ci dirà qualcosa di più.

ulteriore, aggiungo io, arretramento del potere d'acquisto delle retribuzioni. Come infatti abbiamo detto tante volte, siamo fermi da trent'anni, anzi facciamo qualche passetto indietro, e nel 2023 passi passi avanti non ne abbiamo fatti: siamo ancora fermi. Si vede qualche barlume di speranza per il 2024 sui rinnovi dei contratti, ma, per stessa ammissione dei rappresentanti dell'Istat, per recuperare il potere d'acquisto perso dagli stipendi dei cittadini italiani quello che dovrebbe essere il primo obiettivo del Governo, se pensasse ai cittadini e non a qualcun altro - ci vorranno molti anni, che non sono stati meglio quantificati. Chissà perché noi chiedevamo l'introduzione di un salario minimo; forse perché avevamo percepito che c'era qualche problema. Non basta l'allarme presentato dall'Istat: vediamo che

centinaia di migliaia di lavoratori in difficoltà, impedendo la proroga di questo provvedimento e fregandovene delle famiglie ancora una volta. *(Applausi)*. Vi riempite la bocca di maternità, natalità, sostegno, però nei fatti non fate fate niente, anzi cancellate anche le misure di chi aveva avuto un occhio più attento di voi per i cittadini. Oltre a ciò, emerge ancora di più l'enorme divario rispetto agli altri Paesi europei sulla condizione femminile, ancora una volta nella conciliazione dei tempi lavoro-vita privata e udite udite - sul benessere economico. Chissà perché abbiamo donne più formate e più istruite degli uomini, ma vengono peggio pagate. Poi si dice che non siamo in una società patriarcale; ma no, figuriamoci, ma dove mai? Ma che film avete visto? Noi lo abbiamo visto bene il film, voi invece ne volete raccontare un altro ai cittadini di questo Paese. Un altro film che raccontate, un'altra fantasia è quella sui conti della sanità, perché l'allarme l'ha suonato, sempre in audizione, la Corte dei conti, che ha evidenziato come l'aumento fittizio, solo a numeri, del Fondo sanitario nazionale, in realtà non tiene il passo con l'aumento dell'inflazione. Capisco che siano concetti forse un po' complessi per chi guarda solo una cifra assoluta e non fa il paragone con il costo della vita - un difetto che abbiamo già evidenziato in questa maggioranza anche per quanto riguarda le retribuzioni - ma l'allarme sui conti della sanità è evidente, tant'è vero che, qui sì, il Ministro ha risposto e non si è nascosto, parlando limpidamente di razionalizzazione dell'offerta sanitaria. Traduco per chi magari non capisce bene che cosa voglia dire: vuol dire tagli; vuol dire che, invece di erogare i nuovi LEA, andiamo ancora a restringere, nelle idee del nostro Ministro dell'economia, le prestazioni ai cittadini. Non è un caso forse che l'aggiornamento dei nuovi LEA, che doveva entrare in vigore dal 1° aprile, è stato rimandato al 1° gennaio gennaio 2025. Tanto i cittadini aspettano quelle prestazioni solo dal 2017, quindi che sarà mai un altro anno di ritardo? Tanto già in 4 milioni hanno rinunciato alle cure; se ne aggiungiamo qualche altro milioncino tanto a voi interessa solo far quadrare i conti, mentre della salute dei cittadini non ve ne frega niente. Siete miopi anche per quanto riguarda i conti, perché tutto quello che investiamo in sanità ha un moltiplicatore quasi di due volte. Quindi, se noi aumentassimo gli investimenti in sanità, faremmo aumentare anche il PIL del nostro Paese. Voi, però, non siete proprio capaci di guardare alla crescita; siete solo capaci di tagliare e il primo taglio ce lo aspettiamo sulla sanità. D'altronde l'abbiamo già visto nel 2023, quando dicevate che stavate aumentando. Invece, a conti fatti, alla fine dell'anno nel 2023 per la salute dei cittadini italiani abbiamo speso meno nel 2022. Voi continuate a dire che non è vero che non state investendo abbastanza in sanità. Quando ammetterete che c'è un problema, forse tutti insieme troveremo il modo per risolverlo. Finché lo negate, state solo facendo del male al Paese e ai nostri cittadini. Vengo al tema centrale di questa giornata di discussione, che è l'enorme spreco fatto con il superbonus in questo Paese. Mi dispiace anche per le parole che ho udito prima dal dal senatore Monti. Certo, perché il superbonus ha fatto disastri: infatti ha fatto crescere il PIL del 13 per cento in due anni, assorbendo i problemi causati dalla pandemia e dandoci una spinta ulteriore, che ci ha fatto balzare ai primi posti per crescita in Europa. Cosa che non si era mai vista perché con le politiche di *austerity* non siamo mai andati da nessuna parte, non abbiamo mai promosso la crescita del Paese e non abbiamo mai ridotto il debito pubblico; siamo solo arretrati. Invece con le nostre politiche abbiamo fatto dei balzi in avanti: 140 miliardi di entrate fiscali aggiuntive, a fronte di soli 41 miliardi di uscite per i crediti fiscali. E la cessione dei crediti, che tanto non piace al Ministro (perché chissà chi vuole favorire), era l'unica misura che aveva aiutato le fasce più deboli della popolazione, quelle che non hanno capienza fiscale, quelle che non hanno soldi in banca da poter spendere per certi investimenti. Raccontiamola nella realtà la storia e non come piace a voi. Vado a concludere, Presidente. L'incapacità totale di questo Governo è evidente a tutti, anche a coloro che la scrivono chiaramente nel DEF, dove dicono che ci sarà una crescita striminzita del solo uno per cento, di cui il 90 per cento è frutto del PNRR. Quel PNRR che, se esiste, è solo merito del presidente Giuseppe Conte, del MoVimento 5 Stelle e della maggioranza che lo sosteneva in quel momento. *(Applausi)*. Ritengo che l'unico risultato certo conseguito da questo Governo e da questa maggioranza sia la conferma che l'Italia è un contraente inaffidabile per i suoi stessi concittadini, per l'Europa e per eventuali investitori stranieri. È conclamata la vostra incapacità di rilanciare la crescita e il vostro totale asservimento alle politiche di *austerity*, che favoriscono chissà chi, ma di sicuro non i cittadini italiani. Questo si evince chiaramente dalla vostra scommessa nascosta all'interno dei dati di questo DEF. *(Richiami del Presidente).* Mi avvio a concludere, Presidente. La non pagabilità dei crediti del superbonus è quello su cui scommettete. Siete incapaci persino di mettere a terra le risorse del PNRR e scommettete sulle mancate uscite che lasciano a carico di cittadini e imprese i costi

Presidente e colleghi, mi permetto innanzitutto di rivolgere un ringraziamento al ministro Giorgetti, che - come è già stato ricordato questa mattina

un ritorno importante a chi lavora per permettere a questa Assemblea e ai nostri cittadini di conoscere il lavoro certosino, che è stato fatto sicuramente da tutto il MEF. Il periodo che stiamo attraversando - come è già stato ricordato - non è sicuramente facile ed è contraddistinto dalle incertezze. Chi non ammette questo è chiaramente in malafede, perché è evidente a tutti il periodo che stiamo vivendo, caratterizzato sia dalla situazione che dagli strascichi che la pandemia Covid ha lasciato nel nostro Paese. Va ricordato che proprio nel periodo pandemico il Patto di stabilità è stato sospeso e che ci stiamo avviando verso un nuovo periodo, in cui entreranno in vigore le nuove regole della *governance* europea. Quest'anno, in via transitoria, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma saranno sostituiti dal Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine; dovrà essere presentato alle autorità europee entro il 20 settembre. Nel corso dell'estate avremo modo di valutare il quadro programmatico; quindi non è vero che è saltato il quadro programmatico, in verrà discusso dopo che sarà stato aggiornato alle nuove regole europee. L'anno 2023 è stato caratterizzato dalla situazione geopolitica che l'ha segnato. La guerra Ucraina e Russia, le tensioni tra Israele e Palestina, gli attriti sul Mar Rosso, i forti incrementi dei prezzi energetici e delle materie prime, il carrello spesa, la forte inflazione e il forte costo del denaro hanno inciso fortemente sull'economia reale del Paese. La resilienza delle nostre aziende e le misure messe in campo da questo Governo hanno permesso di sostenere i consumi delle famiglie, soprattutto le fasce deboli. Credo sia importante ricordare che, proprio nel corso del 2023, il taglio del cuneo fiscale previsto nella legge di bilancio è stato incrementato a maggio con un investimento pari a 10 miliardi di euro. Abbiamo consentito di mantenere il potere d'acquisto alle famiglie e alle fasce deboli, quelle che voi spesso dite di difendere, ma solo a parole. C'è voluto il Governo di centrodestra per sostenere le famiglie. Il 2023 è stato anche caratterizzato da un aumento del tasso di occupazione rispetto al 2022, incrementato di

Questi elementi sono quelli che sosterranno il consumo nei prossimi mesi. Gli investimenti beneficeranno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e speriamo presto nell'allentamento della politica monetaria che, se non erro, dalle informazioni che abbiamo, dovrebbe avvenire nel mese di giugno. Noi lo auspichiamo perché ciò ha veramente messo in difficoltà tante famiglie e tante persone che hanno i mutui sulle spalle.

evidentemente gli effetti del *bonus* edilizio. Ricordo in quest'Aula che questa misura è costata 219,5 miliardi, con un beneficio sugli immobili

Presidente, credo che il Governo di centrodestra abbia ereditato una situazione non semplice da gestire, non solo per il delicato momento di tensioni geopolitiche che stiamo attraversando, ma anche per le misure scellerate messe in campo dai Governi precedenti (ringrazio il senatore Monti per aver ricordato alle opposizioni che hanno influito sulla situazione attuale) che gravano sui bilanci dello Stato e, di conseguenza, sui cittadini. Ho già citato la misura del *superbonus*, che è un'eredità pesante, ma non vanno dimenticate nemmeno misure come il reddito di cittadinanza (che ha creato non occupazione, ma solo mancanza di manodopera all'interno delle nostre aziende) o i famosi banchi a rotelle, di cui ancora oggi

sui dispositivi medici, penalizzando quel settore d'eccellenza e di ricerca, ha creato ingenti costi.

le sfide che abbiamo davanti non sono facili, la linea che questo Governo ha assunto va nella direzione corretta e, nonostante tutte le difficoltà che incontriamo sul nostro percorso, dovute a fenomeni esterni o a scelte precedenti, non viene meno il sostegno che gli elettori hanno manifestato verso questa maggioranza. La Lega c'è e continua a lavorare perché il Paese sia forte e possa essere competitivo negli anni a venire nell'Europa che sarà. *(Applausi)*. Signora Presidente, Sottosegretario, colleghi, esiste una profonda contraddizione tra un quadro macroeconomico certamente complesso, per non dire drammatico, nel quale le relazioni internazionali sono messe a dura prova da tensioni e conflitti insorti in molte aree del mondo (pensate che le Nazioni Unite individuano nel 2023 l'anno con il maggior numero di conflitti dopo la Seconda guerra mondiale)

di una bussola, di una visione, di una capacità di programmazione che oggi sarebbe ancora più importante, a fronte di un quadro macroeconomico così complesso.

solo Governi dimissionari o che stavano per esaurire il proprio mandato non presentavano il documento programmatico. Siamo in presenza, dunque, di una discussione di basso profilo che a mio avviso rappresenta un fallimento da parte di questo Governo sulle politiche economiche e sociali, perché anche di fronte alla nuova *governance* europea è necessario rispondere con una visione economica, economica, con un profilo programmatico, non con un rinvio che ha solo lo scopo di tirare a campare, di far passare le elezioni senza nessuno sguardo al futuro di questo Paese e dunque alle future generazioni. Questo è un vostro fallimento *(Applausi)*. Lo dico perché purtroppo la frammentazione dell'economia globale dentro questi conflitti tra blocchi sempre più contrapposti espone a conseguenze importanti, difficili e perfino drammatiche anche l'Europa. Sappiamo tutti che c'è una stretta integrazione produttiva e finanziaria tra l'Europa e il resto del mondo. Sappiamo tutti che il nostro modello di sviluppo dipende dall'importazione di risorse naturali. Sappiamo tutti che senza una visione, nel tirare a campare, nel trovare i colpevoli, l'Europa rischia di indebolirsi.

assente nella costruzione di una nuova Europa. Senza politiche economiche e sociali, la nuova Europa non nasce. Mi rivolgo ai colleghi di Fratelli d'Italia: ricordatevi che siete al Governo Governo e ai colleghi della Lega ricordo che hanno governato anche di fronte ad una fase difficile post-pandemica nella legislatura precedente dunque non basterà la continua retorica del fare opposizione all'indietro. *(Applausi)*. Oggi serve un futuro a questo Paese e i Governi sono chiamati ad indicare una rotta e dovreste anche essere nelle condizioni di mettere l'opposizione, dunque questo Parlamento, un'altra volta nella dimensione centrale che la Costituzione gli assegna. Ora, diciamocelo con grande franchezza: siamo in presenza di un Governo senza una bussola. Questo DEF è il vostro fallimento e non viola solo una legge importante, approvata in questo Parlamento, cioè la legge di contabilità. Presidente, normalmente (io credo che sia un principio da ristabilire) si può modificare una legge, ma finché non la si modifica o finché non si aprono le procedure per modificarla, la si rispetta. Sono regole costituzionali già previste nel nostro ordinamento, mentre in questo caso siamo in presenza di una violazione senza l'apertura di nessun confronto tra maggioranza e opposizione su uno dei terreni più importanti, che sono le regole contabili, le norme che regolano i saldi di finanza pubblica. Io sono molto preoccupato della deriva che sta assumendo anche il Ministero dell'economia e delle finanze, perché di fronte a questo quadro così incerto vedo tentazioni tricefale,

Vedo chi sta indicando una presunta riforma fiscale epocale, che invece rappresenterà non solo il consolidamento in negativo dell'attuale assetto, che rappresenterà per i prossimi anni anche un elemento di ulteriore incertezza sulle entrate, perché attraverso l'introduzione di condoni e di meccanismi fiscali che chiamate sotto falso nome, ma che in realtà incentiveranno nei prossimi anni più elusione e più evasione, state anche realizzando un carico fiscale insostenibile nei confronti di chi paga l'IRPEF. State anche producendo vantaggi fiscali per il lavoro autonomo. Ricordiamoci che per noi le partite IVA sono un elemento fondamentale in questo Paese: sono lavoro, innovazione, possibilità di intraprendere la strada del promuovere un'impresa, non c'è alcun dubbio. Tuttavia i parametri fiscali ormai lasciano il 47 per cento della pressione fiscale sul lavoro dipendente e su chi paga l'IRPEF, mentre abbiamo introdotto meccanismi del 15 per cento di tassazione piatta favorevole; l'Italia è il Paese in Europa con più lavoro autonomo, tre volte rispetto agli Stati Uniti. Dove vogliamo andare? Altro che riforma epocale; è una riforma che nei prossimi anni, purtroppo, indebolirà anche le buone e corrette politiche di riforma del sistema fiscale che avevamo introdotto, soprattutto nei confronti della digitalizzazione della riscossione, dell'informatizzazione della stessa, di una vera e importante lotta all'evasione fiscale che abbiamo costruito negli anni precedenti. State smantellando il sistema fiscale addirittura con l'ideologia del "meno tasse per tutti", quando sapete bene che tale retorica non è compatibile con l'attuale quadro di finanza pubblica. Se aggiungo anche che si sta mettendo in discussione la neutralità, il ruolo importante della Ragioneria generale dello Stato, anche chi si ispira ad antiche visioni keynesiane dell'economia deve ricordarvi con grande franchezza che è importante, all'interno di una dinamica così delicata, la solidità del processo culturale e politico che il Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria dello Stato negli anni hanno sempre saputo salvaguardare. Questo, infatti, è il terreno della democrazia, non dell'uomo solo al comando, o, peggio ancora, di una situazione nella quale il Parlamento è costretto ad essere ai margini delle dinamiche di trasformazione e di riordino. Diciamoci con grande forza e serenità tra di noi in quest'Aula che non c'è una proposta. L'unico documento presentato dall'Ufficio parlamentare di bilancio che simula quello che potrà accadere dentro la nuova *governance* europea rende l'Italia più sola, più debole in Europa, oggi anche meno credibile per quello che siete riusciti a rappresentare in Europa anche ieri. Infatti non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo: il Ministro dell'economia in quest'Aula ha detto con chiarezza che la mediazione costruita sul nuovo Patto di stabilità È venuto in questa sede a promuovere l'accordo, quando tutti noi avevamo sempre ritenuto che fosse preferibile sostenere per intero, dentro alleanze europeiste e non nazionaliste, la proposta del commissario commissario Gentiloni *(Applausi)*, che era sicuramente più flessibile nelle relazioni, ovviamente anche con la gestione di uno dei pezzi più pregiati e difficili che abbiamo da difendere, che è la collocazione del nostro debito. Voi non siete preoccupati di un debito che cresce, ma ci sono i dati, i numeri. E non siete nemmeno preoccupati di un ritorno allo zero virgola della crescita, perché sappiamo tutti che in economia l'unico sentiero per una gestione ordinata del debito è una crescita economica. Dovreste venire in quest'Aula con un'agenda delle riforme diversa da quella che state impostando; cambiatela in fretta. Ci fate discutere di autonomie differenziate e di premierato, quando occorrerebbe rivedere i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, ispirandoci ad una cooperazione istituzionale e non ad una contrapposizione. State producendo le riforme che non servono, ovvero che servono solo a voi, per la gestione del potere, mentre non servono alle famiglie e alle imprese italiane per avere più servizi, più diritti, più equità e più giustizia sociale in questo Paese. Portate la riforma della sanità in quest'Aula, se volete affrontare uno dei perni fondamentali dei diritti di cittadinanza, che si stanno già negando. Portate una riforma strutturale dei sistemi di istruzione e di formazione, perché il futuro di questo Paese passerà attraverso la formazione delle risorse umane. Portate in quest'Aula una riforma per garantire il salario minimo e per affrontare uno dei problemi più importanti che abbiamo di fronte: bassi salari e bassa produttività. dello sviluppo economico, se non sostenete la transizione ambientale, digitale e sociale, che è l'unica leva fondamentale per salvaguardare una nuova manifattura e una nuova capacità produttiva, voi rischiate che non solo tutta l'Europa, ma anche l'Italia, diventi un mercato e non più un luogo produttivo per generare futuro e speranza per le giovani generazioni. Cambiate l'agenda delle riforme.

del Governo, colleghi, oggi ci accingiamo ad analizzare ed esaminare l'ultima versione nel modello classico, che c'è sempre appartenuto, del Documento di economia e finanza. in quanto, come sapete, l'Unione europea lo sostituirà con il Piano fiscale-strutturale di medio termine e con il Rapporto di monitoraggio annuale. Questo DEF, ovviamente, è stato disegnato anche guardando quali sono gli scenari internazionali che purtroppo colpiscono ogni giorno l'Europa, l'Italia ed i mercati. Sono scenari non del tutto gradevoli e favorevoli all'economia, anche se c'è da dire che l'economia mondiale e le condizioni finanziarie vedevano dei miglioramenti soprattutto rispetto alla vecchia NaDEF. La nostra economia, come giustamente ha ricordato il ministro Giorgetti, si è sempre distinta per un grado di resilienza a fronte dei continui *shock* che, purtroppo, subiamo costantemente negli ultimi anni. La crescita dell'occupazione, per fortuna, è in continua ascesa ed anche il dinamismo del PIL ha degli aspetti migliorativi. Come dicevo, le tensioni internazionali, da ultimo

rischiano veramente di determinare per il nostro Paese delle condizioni economiche difficili. Ciò soprattutto per quanto riguarda il sistema delle esportazioni e anche delle importazioni delle merci che arrivano e devono passare attraverso il canale di Suez. Ciononostante, l'economia italiana sta dimostrando grande resilienza, sebbene questa instabilità politica sia continua e persistente. Il quadro macroeconomico, ovviamente, è debole e induce a prevedere margini di crescita, utilizzando spazi finanziari per ridurre il cuneo fiscale ed andando avanti con le riforme fiscali già annunciate e promesse dal Governo. Banca d'Italia descrive positivamente gli andamenti macroeconomici delineati nel DEF, sostenendo che le stime del Governo non sono differenti dalle loro previsioni aggiungendo che, nel complesso, siano ricomprese nel ventaglio delle proiezioni dei principali previsori, collocandosi tra quelli più positivi. Aggiungo poi che anche le stime dell'Istat confermano una crescita occupazionale, a febbraio, di altre 41.000 unità. Una crescita, quindi, dovuta all'aumento dei dipendenti permanenti, che sfiora i sedici milioni di unità. Allo stato attuale, il numero di occupati nella nostra Nazione equivale a 23.773.000 unità, superando di ben 351.000 unità il numero di occupati dello scorso anno, con un aumento dunque significativo. Il tasso di occupazione è a livelli *record* (61.9 per cento) e rappresenta un altro tassello del mosaico vincente che il Governo Meloni sta dimostrando non solo nel Paese, ma anche e soprattutto in ambito internazionale. non lo diciamo noi, poiché non sono le solite prese di posizione della nostra parte politica; sono dati, numeri che provengono da un organismo internazionale *super partes* quale l'OCSE, che fotografa gli ultimi anni degli indicatori economici del lavoro in Italia. Ebbene, l'OCSE conferma come l'Italia sia tra i Paesi che hanno segnato le *performance* migliori a fine 2023. L'agenzia Standard & Poor's conferma il nostro *rating* - e questo è positivo - nonostante lo scenario, come dicevo prima, particolarmente complicato. Il «New York Times», come larga parte della stampa straniera, specie e soprattutto quella anglosassone, e nell'ultimo periodo devo dire anche «Le Figaro» (quindi anche la stampa francese) hanno espresso giudizi complessivi positivi nei riguardi del Governo italiano, in particolare nei confronti del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. La rivista statunitense «Time» loda la nostra *Premier*, sostenendo che quando la *Premier*, la prima donna italiana a diventare Presidente del Consiglio, è salita al potere nel 2022, molti osservatori nutrivano dei timori per l'impatto che avrebbe avuto sull'Italia, sull'Europa e sul mondo. Ma a due anni di distanza la presidente Meloni rimane popolare non solo in Italia, ma anche tra i *leader* occidentali, molti dei quali si sono rallegrati del suo fermo sostegno all'Ucraina e per la diplomazia in ambito internazionale, sicura e affidabile, che ha contraddistinto il suo operato. Non dimentichiamoci poi dello *spread*, che mai è stato così basso come in questo periodo: il differenziale di rendimento fra titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è ai minimi dal 2022, merito certamente del Tesoro, che colloca i titoli di Stato, ma anche e soprattutto dell'azione del Governo, la cui serietà e il rigore dimostrati sono stati apprezzati dai mercati finanziari e dagli investitori internazionali. La particolare attenzione ai mercati internazionali rassicura la politica estera. Cito inoltre gli interventi di sostegno e di politica economica e sociale per fronteggiare, in particolare, l'emergenza energetica e la riforma fiscale, che ha profondamente ridisegnato l'intero sistema tributario, ammodernandolo come non accadeva da decenni e accrescendo la credibilità del Paese agli occhi degli investitori nazionali ed esteri. sono solo alcuni temi relativi ai traguardi di cui siamo particolarmente orgogliosi, sebbene una sinistra catastrofista continui goffamente a disconoscerli. Gli interventi normativi, come quelli che dicevo poc'anzi, introdotti a partire dall'inizio di questa legislatura, sono apprezzati dagli italiani e dai mercati finanziari, ed hanno un impatto sul tessuto socioeconomico italiano positivo e durevole. Soprattutto, essi fondati sul realismo, in un contesto internazionale che permane certamente complesso e preoccupante per tutti, non solo per la nostra Nazione. Dopo l'attacco dell'Iran a Israele, i rischi di potenziali danni correlati relativamente al Mar Rosso rimangono elevati, anzi aumentano. Le conseguenze economiche per l'Italia, già di per sé gravi, dallo scorso gennaio rischiano infatti di essere davvero sfavorevoli e dannose, considerato che la crisi costa all'*export* italiano 95 milioni di euro al giorno, per un totale di 8,8 miliardi di euro di danni, a causa dell'impatto del calo di traffico di navi mercantili dall'Oceano Indiano al Mar Rosso, come dicevo prima. La guerra purtroppo ancora in corso tra la Russia e l'Ucraina e altre situazioni di conflitto che continuano a sorgere in diverse parti del mondo hanno inciso in maniera evidente nella programmazione degli aggregati macroeconomici e di finanza pubblica e, di conseguenza, nelle decisioni della politica economica del Governo, rivedendo le stime di crescita e gli investimenti. Vi è poi un capitolo a parte che ha condizionato pesantemente il DEF per il 2024, quello relativo al superbonus. pubblici, come è noto, pesa l'impatto della zavorra del superbonus, arrivato al capolinea lo scorso 4 aprile, con lo stop deciso dal Governo con un decreto *ad hoc*, anche per la remissione *in bonis*. Al momento, il complesso dei *bonus* edilizi ha portato il *deficit* per il 2023 al 7,2 per cento, contro il 5,3 stimato nell'autunno scorso dall'Istat. Senza la fiducia dei risparmiatori italiani e della comunità internazionale risulta difficile non solo immaginare un nuovo debito buono, ma anche la gestione del vecchio debito che abbiamo ereditato. È un'eredità pesantissima per i conti pubblici e quindi per tutti gli italiani, della cui realtà nei prossimi anni dovremo farci carico per pagare il debito pubblico in risalita (che rimane tuttavia sotto la soglia del 140 per cento), che è stato fatto grazie alle politiche assurde, scellerate e assistenzialiste dei Governi Conte, che hanno determinato un impatto devastante di 219 miliardi di euro causati dai *bonus* edilizi. Aggiungo che le comunicazioni piovute dall'Agenzia delle entrate per certificare gli sconti e le cessioni in fattura dei *bonus* edilizi del 2023 hanno creato un'altra onda in piena della spesa, con una trentina di miliardi aggiuntivi rispetto a quelli che già conoscevamo. Vale la pena ricordare che lo scorso anno si è deciso di finanziare la manovra economica per il 2024 aumentando il *deficit* programmatico della NADEF di 0,7 punti rispetto al tendenziale della Nota di aggiornamento, proprio proprio a causa degli effetti che il superbonus aveva determinato sui saldi di finanza pubblica. Pertanto il compito principale del Governo nell'elaborazione di questo DEF è stato giustamente - e aggiungo responsabilmente - quello di mettere un punto fermo ad una finanza pubblica sull'altalena a causa dei crediti di imposta, che hanno un impatto pesante sulla crescita, sull'indebitamento e sul *deficit*. In questo contesto, il Documento di economia e finanza che ci accingiamo a votare risponde alle esigenze, comuni agli altri Paesi membri, di tenere conto della rivoluzione delle regole che l'Unione europea ci impone. Le previsioni programmatiche annesse di eventuali spese e/o correzioni arrivano con il Piano strutturale da presentare entro il 20 settembre, che rappresenterà la cornice della manovra 2025. Nel Documento economico la crescita del PIL a legislazione vigente è pari all'1 per cento per quest'anno e all'1,1 per cento per il prossimo; stime confortate anche da Confindustria. Il sostegno ai redditi dei lavoratori, avvenuto prevalentemente, ma non solo, tramite la riduzione contributiva, ha consentito anche di moderare la spinta salariale...

festeggiare, il prossimo 1° maggio, la festa dei lavoratori. Credo che in questo 1° maggio sia giusto anche ricordare quanto fatto dal Governo Meloni Meloni nei confronti della diminuzione del cuneo fiscale, perché questo i lavoratori italiani lo stanno sentendo nelle loro buste paga. L'obiettivo del

l'affetto e l'amicizia che abbiamo (si può essere avversari politici, ma continuare a essere amici), ma soprattutto perché abbiamo fatto parte di uno stesso Governo. Io mi metto quindi nei suoi panni, anche perché lei ama come me la musica classica ed è persona di grande cultura, mi metto nei suoi panni elegantissimi

Dai banchi dell'opposizione, oggi attuale maggioranza, si diceva che quei numeri erano un mero rimbalzo perché avevamo avuto una pandemia più drammatica rispetto all'Europa e che non corrispondevano a una crescita economica vera, come succede nei momenti di grande crisi.

0,3. Quando si governa bisogna essere esaltati da numeri che non sono esaltanti non solo perché non permettono di realizzare quel libro dei sogni della riduzione delle tasse che avete offerto agli italiani durante la campagna elettorale, ma perché non servono a risolvere i problemi esistenti in questo Paese. Anzitutto, una crescita economica non soddisfacente impedisce di fare quegli investimenti che avrebbero dovuto essere realizzati dal PNRR e che in parte avete anche restituito all'Europa. Le categorie economiche sono quindi molto preoccupate. Ad esempio, una legge fondamentale per l'imprenditoria è la nuova Sabatini, che ogni anno sembra non essere rinnovata. Eppure da quella legge gli imprenditori che vogliono investire nel nostro Paese ricevono una linfa vitale. Vogliamo parlare del mondo agricolo? Siamo passati dall'aver rimesso l'IRPEF agli agricoltori all'averla tolta in parte, ma soprattutto aver messo delle tasse, come

Soprattutto, in un mondo che cambia velocemente e dove noi dobbiamo competere non soltanto col nostro vicino francese, austriaco e spagnolo, ma con il mondo intero, non investire risorse risorse affinché la nostra industria e il nostro modo di fare impresa possano essere adeguatamente sviluppati è un male che facciamo a noi stessi. E invece pare che il Ministero che una volta si chiamava dello sviluppo economico e che adesso si chiama delle imprese e del *made in Italy* sia più preoccupato dal nome di un'auto, che non da come produrre quell'auto nel nostro Paese. Paese. Da torinese posso dire noi abbiamo sempre una certa competizione con Milano, ma il gusto di vedere la parola Milano nell'Alfa Romeo non mi turbava. Forse mi turba molto di più la parola *junior,* perché mi sembra di vivere in un mondo non mi pare abbastanza bizzarro che, rispetto a un nome italiano, si sia preferito un nome anglofono da parte di chi diceva invece di voler togliere qualsiasi riferimento straniero nelle leggi italiane. Da torinese dico che la preoccupazione della città di Torino è se Stellantis, *ex* FCA, *ex* FIAT, continueranno a produrre nel nostro Paese, con che dimensioni e capacità. e capacità. Se leggo le dichiarazioni dei Ministri scopro, per esempio, che il ministro Pichetto Fratin ha deciso di far produrre reattori nucleari a Mirafiori. Avendo prodotto le mascherine durante la pandemia, che da servizi giornalistici sono apparse neanche troppo ben fatte, non vorrei che i reattori nucleari fatti da una fabbrica che in realtà dovrebbe fare automobili provocassero incidenti disastrosi. Piuttosto di fantasia al potere, cerchiamo di capire come investire le risorse che il PNRR, per esempio, ha fornito per la transizione ecologica proprio in una realtà che non si è rassegnata a non avere quella fabbrica nella propria città. Non mi riferisco solo alla città di Torino, perché sappiamo che l'*ex* FIAT, oggi Stellantis, è in tutta Italia e ci sono lavoratori preoccupati. preoccupati. Il 1° maggio si va in piazza a dire: evviva, il Governo Meloni ha fatto tanto per i lavoratori. Ma, partendo dalle risposte date alle imprese e alla produzione in Italia, si riuscirebbe forse a dare più credibilità a questa frase e anche a questa festa. festa. Signor Sottosegretario, penso che il libro dei sogni sia una cosa molto bella, ma la realizzazione di questi sogni, in questo DEF, non c'è. Eravamo pronti, lo scorso anno, a sentir dire: d'altronde non l'abbiamo scritto noi, siamo appena arrivati e quindi dovete lasciarci fare e darci un po' di tempo per governare, vedrete il prossimo anno cosa succederà. Ebbene, era questo l'anno in cui si doveva vedere che cosa sarebbe successo e non è successo assolutamente niente. Concludo col dire che le preoccupazioni del mondo produttivo dovute alle incertezze della geopolitica, ma anche ad un'incertezza, ad una visione economica di questo Paese, creano un turbamento molto più forte di quanto forse le dichiarazioni di qualche presidente compiacente di qualche categoria dicano, perché quando si va nel cuore del Paese,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, lo hanno detto molti miei colleghi prima di me, ma lo voglio sottolineare anch'io: questo DEF, che il Governo annuncia essere stato redatto in forma semplificata, in realtà è vuoto perché è vuota la vostra azione di Governo, che non ha una strategia per l'Italia. È vuoto perché è vuota la vostra impostazione, perché se da un lato le previsioni confermano un progressivo calo del rapporto fra spesa e PIL, non si possono escludere ulteriori tagli rigorosamente da fare, ovviamente, solo e soltanto dopo le elezioni europee e che oggi nascondete, anche perché basta guardare quanto sono risicati i margini per finanziare in *deficit* la prossima manovra. E allora, se sarà necessario, cosa andrà a tagliare il Governo? Noi temiamo che sarà tagliata ulteriormente la sanità. ulteriormente, Presidente, perché a differenza di quanto si affanna a ripetere il Governo, e cioè di avere ottenuto il *record* di finanziamento della sanità, è vero il contrario.

la spesa sanitaria rispetto al PIL era al 6,3 per cento nel 2023, scenderà al 6,2 tra il 2025 e il 2027. direte di non guardare la spesa rispetto al PIL, di parlare solo di valori assoluti. Bene, allora parliamo di quant'è la stata la spesa sanitaria nel 2023: 131 miliardi, 3,6 miliardi in meno rispetto al 2022. Queste bugie, Presidente, stanno già diventando un *boomerang*. Pensate che non se ne accorgano, i cittadini italiani, che state smantellando il Servizio sanitario nazionale pubblico e universale? Basta andare al bar, Proprio ieri un mio vicino di casa mi ha raccontato che per operarsi di un'ernia avrebbe dovuto attendere un anno e mezzo e si è rivolto alla sanità privata; lui può permetterselo, ma chi non può sta rinunciando a curarsi. Lo sapete che nella stragrande maggioranza degli ospedali d'Italia a settembre finiscono le protesi di anca? Chi si rompe il femore dopo questa data deve aspettare a gennaio dell'anno successivo per operarsi. Queste cose i cittadini italiani le vedono e non credono alle vostre bugie, ma se non volete ascoltare il grido d'allarme che lanciamo noi da questi banchi e che lanciano i cittadini italiani, se li incontraste per strada, allora potreste ascoltare l'appello degli scienziati, dei medici, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi dello scorso 3 aprile. Questi eminenti cittadini partono dalla considerazione che dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 in Italia il Servizio sanitario nazionale ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell'aspettativa di vita: siamo passati da 73,8 anni a 83,6 anni tra i Paesi ad alto reddito. I dati però dimostrano che il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle disuguaglianze regionali Questo accade perché - dicono gli scienziati - i costi dell'evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e le difficoltà della finanza pubblica hanno reso fortemente sottofinanziato il Servizio sanitario nazionale, al quale nel 2025 sarà destinato il 6,2 per cento del PIL, cioè meno di vent'anni fa.

ha detto: non mettiamo in discussione una difesa della vita delle persone così attenta ed importante come la sanità pubblica; il nostro Servizio sanitario nazionale deve rimanere una garanzia fondamentale per tutti e di tutti. Lo ha dichiarato solo due giorni fa. Tuttavia, se non volete ascoltare neanche monsignor Zuppi, allora potreste ascoltare la Corte dei conti, che, in audizione sul DEF, ha certificato una condizione deficitaria per la sanità pubblica ed il fallimento delle politiche adottate. la Corte dei conti emerge un quadro di una situazione in decadimento del Servizio sanitario nazionale, che dovrebbe vedere maggiori finanziamenti. finanziamenti. Aggiungo che servono risorse per il taglio delle liste di attesa, per l'assunzione degli operatori sanitari, per le reti di assistenza territoriale, giusto per fare qualche esempio. Avviandomi a concludere il mio intervento, le colleghe e i colleghi di maggioranza non volessero ascoltare i cittadini italiani, noi del Partito Democratico, gli scienziati, la Chiesa, la Corte dei conti, allora possono avventurarsi a dire che va tutto bene, ma saranno i cittadini italiani a tapparsi le orecchie e non credere più alle loro fanfare. Signor Presidente, signor Sottosegretario, comincio subito col dire che il presente Documento di economia e finanza è inadeguato alla fase che stiamo attraversando. Siamo consapevoli e sono consapevole, ad esempio, delle difficoltà e del rischio di incidere negativamente rispetto alla situazione generale data dalle guerre, dal rialzo dell'inflazione, eccetera. Tuttavia, il DEF in esame,

una scelta di questo tipo la fanno i Governi tecnici o i Governi dimissionari. Mi viene un dubbio, però, perché ieri è successo un fatto significativo Il ministro Giorgetti è venuto in audizione e ci ha spiegato che lui a nome del Governo aveva concordato sulla *governance* europea un accordo,

non tecnico ma dimissionario, oppure dovete spiegarmi come si deve fare. Io sono d'accordo sul fatto che non dobbiamo accettare di ritornare all'austerità,

DEF è affidarvi alla questione di sostenere la domanda attraverso il cuneo fiscale e non c'è alcun intervento su questioni importanti come, ad esempio, la limitazione dei prezzi. La benzina ormai è oltre i 2 euro

la condizione materiale delle persone che lavorano e dei pensionati, oltre a quelli disagiati, sta peggiorando. In tutto questo non fate una cosa: andare a prendere i soldi là dove ci sono. Fate una manovra restrittiva, restrittiva, indicate una tendenza di bilancio molto restrittiva e - una cosa è chiara - non andate a prendere i soldi attraverso la tassazione delle rendite finanziarie

Abbiamo parlato di eroi, di persone che hanno risposto in prima persona di fronte alla pandemia, però il contratto è scaduto, quello rinnovato è scaduto nel 2021 e adesso prevedete solo l'indennità di vacanza contrattuale. Non c'è un piano di occupazione pubblica per rispondere all'elevato numero da una parte di pensionamenti, dall'altro per rafforzare e riqualificare il sistema pubblico. Questo è un dato fondamentale se vogliamo modernizzare questo Paese. Non esiste una politica industriale

alla siderurgia, con tutte le difficoltà che ci sono. Lì ci sono migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici, per non dire milioni, che hanno bisogno, da una parte, di essere sostenuti

fronte a una proposta che non ha una visione complessiva di che cosa bisognerebbe fare. Eppure, noi abbiamo una situazione, da un certo punto di vista, unica, cioè la disponibilità economica dei soldi erogati dal PNRR. In sostanza, quella indicazione significa intervenire sulle disuguaglianze; disuguaglianze che ci sono, da un punto di vista produttivo e da un punto di vista sociale: il riequilibrio tra Nord e Sud, tra il centro e la periferia, tra le zone montane, le zone interne e le città. In sostanza, il progetto dov'è? Questo è il dato che manca. La critica che noi facciamo è una mancanza di visione complessiva da questo punto di vista. In sostanza, voi non intervenite e continuate a non voler affrontare la questione

problema del salario minimo, e, dall'altra, la questione della riduzione dell'orario di lavoro. A fronte del fatto che verranno introdotte nuove tecnologie e di ridistribuzione complessiva; altrimenti, c'è solo qualcuno che guadagna e tutti gli altri che perdono e, allo stesso tempo, come ho già detto ieri, ovviamente c'è anche la paura di fronte al nuovo che dovrebbe avanzare.

le questioni del *welfare*, dei servizi e di incremento delle piante organiche servono risorse strutturali. In questo caso, bisogna andarle a prenderle dalla tassazione. Invece, voi fate dei condoni

si allinea a queste nuove norme, a queste nuove regole, che entreranno in vigore nel prossimo 2025. Già da oggi, però, è iniziato un percorso di aggiustamento ed anche di scrittura di nuovi documenti contabili. È in atto la riforma della *governance* europea, come è anche in atto il nuovo documento riguardante il Piano strutturale di bilancio di medio termine. Quindi, anche i documenti di economia e finanza vengono scritti in maniera differente e siamo in un momento di transizione.

che mantenere e guardare quella che è oggi la fotografia economica reale del nostro Paese. Come dicevo, a breve scriveremo dei nuovi documenti,

Come dicevo, lo vedremo anche prossimamente. Quindi vi è un nuovo sistema, anche di programmazione stessa della spesa, con un monitoraggio molto più attento e un controllo soprattutto della spesa

sono queste oggi le parole chiave di proiezione del DEF e soprattutto degli impegni del Governo in campo economico. Fino ad oggi,

che hanno dimostrato, nonostante una pandemia e tutto quello che abbiamo passato in questo periodo, una grande resilienza. È oggi la forza del nostro Paese. Ecco perché dobbiamo essere al fianco dello sviluppo dell'economia e soprattutto dell'impresa. Se guardiamo gli impegni enunciati nel DEF, restano intatti tutti quelli assunti nel settore della sanità, della trasformazione e della transizione ecologica ed energetica, con la costruzione di infrastrutture molto importanti; una strategia strutturale, per rendere strutturali le politiche importanti per la natalità, per le famiglie e per le donne in particolar modo; tutta una serie di impegni che questo Governo ha intenzione di portare avanti e che mantiene. Poi c'è la battaglia delle battaglie. Siamo arrivati già

fermo questo impegno; come dicevo, gli obiettivi già raggiunti sono i dieci decreti fiscali adottati. Si prevede di rafforzare la coesione territoriale, anche grazie

ha raggiunto per quanto riguarda il numero degli occupati, che oggi vengono associati e implementati in particolar modo alle politiche attive in materia di lavoro, perché serve coinvolgere altri 3 milioni di persone, che devono appunto avere una formazione specifica per entrare nel mondo del

e avere una fotografia reale di quello che accade al Paese. Partendo da questi risultati, partendo da tutto quello che è stato fatto in questo anno e mezzo, partendo dagli obiettivi già raggiunti, il programma del Governo non cambia, nonostante in Europa siano in atto dei cambiamenti che noi guardiamo guardiamo e seguiamo con interesse, insieme a tutti gli altri Paesi europei. Ecco perché noi condividiamo perfettamente oggi quello che andiamo ad approvare con questo Documento di economia e finanza e quindi condividiamo la linea imposta dal Governo.

ad assistere a un nuovo *record* negativo di questo Governo: la prima volta che un Governo con i pieni poteri - come vi piace definirvi - approva un DEF che è solo tendenziale. In genere questo succede per i Governi dimissionari. Voi invece siete nel pieno del vostro mandato e avete però scelto di nascondervi dietro le vostre bugie e di non dire ai cittadini cosa intendete fare nei prossimi anni. Non solo avete i poteri e i titoli per fare un DEF programmatico, ma avete anche il dovere di dire ai cittadini italiani cosa avete in programma per i prossimi anni, quali riforme e quali investimenti. Invece avete deciso di non farlo e di continuare a parlare del passato, perché anche la discussione surreale di oggi, qui e alla Camera, è tutta basata sul superbonus, una misura che - vorrei ricordarlo è stata gestita dal ministro Giorgetti anche nel Governo precedente. Sono tre anni che questo Ministro sta gestendo il superbonus e non mi sembra sia una novità. Se poi nemmeno riesce a classificare i crediti del superbonus, io forse

candidamente dove intende puntare e dove stiamo andando. Il Ministro intende puntare sull'austerità, perché dire che il debito buono non deve diventare debito a tutti i costi vuol dire questo; vuol dire austerità, vuol dire austerità, con tutti i suoi pilastri, con le privatizzazioni selvagge - lo abbiamo visto anche su *asset* strategici - con la precarizzazione del lavoro, con il lavoro povero, povero, con i tagli alla spesa pubblica. Mi vorrei soffermare soprattutto sui tagli alla sanità, per provare una volta per tutte a smascherare le continue bugie del Governo su questo tema. Partiamo come sempre dai dati:

Questi sono i dati che avete scritto voi, nero su bianco: non è l'opposizione a parlare del 6,3 per cento, tanto che "Il Sole 24 Ore" dice che si tratta del tasso di investimento più basso sulla sanità dal 2007.

La seconda bugia è sugli investimenti in termini assoluti, che vi appassionano tanto e sono la vostra ossessione: continuate a dire che invece in termini assoluti stiamo mettendo più risorse. Ma anche questa bugia viene smascherata in questo DEF, in cui c'è scritto che avete speso 131,6 miliardi nel 2022 e 131,1 miliardi nel 2023. Tra 2022 e 2023 quindi, anche in termini assoluti, la spesa è scesa: questi sono i numeri; se poi non sapete leggere quello che scrivete, è un vostro problema. *(Applausi)*. Prevedete un lieve rialzo nel 2024, spostando le risorse che non avete speso nel 2023, per fare il solito gioco delle tre carte a cui ci avete abituato. Del resto, hanno smentito le vostre ricostruzioni tutte le audizioni che sono state fatte, se perfino la Corte dei conti, nel rapporto che ha depositato alle Camere, ha detto che anche nel 2024 quel lieve incremento sulla spesa sanitaria totale non sarà sufficiente a coprire i costi dell'inflazione. Ci sono poi i dati che vanno in parallelo rispetto ai tagli che state operando alla spesa pubblica, in particolare alla sanità: quelli dell'Istat ci dicono che nel 2023 le persone che hanno rinunciato alle cure - perché non possono permettersi la sanità privata e non possono attendere le liste d'attesa, che ormai sono lunghissime - sono passate da 4 a 4,5 milioni. Questa è la fotografia di un Paese che oggi si deve indebitare per accedere a un diritto. *(Applausi)*. L'autonomia differenziata non farà che peggiorare questa situazione, se già oggi ci sono Regioni disagiate in cui la spesa pubblica è più bassa di 4.000 euro *pro capite* per i cittadini che ci vivono. Anche in sanità spendere di meno vuol dire fare meno prevenzione, meno controlli e meno visite specialistiche; dire a un cittadino - come rivelano i dati di Cittadinanzattiva - che deve aspettare due anni per una mammografia o mesi per una visita specialistica vuol dire fargli scoprire di avere un tumore quando ormai non si potrà più curare. Questi sono i dati ed è tutta colpa vostra. *(Applausi. Commenti)*. Lo so, senatore Zaffini, è difficile accettare la verità, ma questo è.

per i bambini autistici, per esempio, partono solamente dopo essere stati in lista d'attesa per due o tre anni, in alcune Regioni, vuol dire di fatto condannare quei bambini a una vita con disabilità. E, quindi, state tradendo l'universalità, l'equità e la giustizia del nostro Servizio sanitario nazionale. Poi ogni tanto provate a dare qualche ricetta e soluzione, che ascolto sempre con grande attenzione:

siamo attenti solo noi a quello che ci dicono tutte le associazioni di categoria in audizione o se ci siete anche voi in quelle aule di Commissione

quei soldi che avevate aggiunto per pagare di più gli straordinari ai medici sono inutilizzati e quindi, se quella è la vostra ricetta per ridurre le liste d'attesa, siamo proprio lontanissimi dalla soluzione del problema. Per ridurre le liste d'attesa ci sono due cose che dovete fare. La prima è assumere personale. Se non ve lo ricordate, c'è ancora quel blocco delle assunzioni di personale sanitario che è stato messo nel 2004 dal Governo Berlusconi È sempre la destra che taglia la spesa sanitaria, è sempre la destra che taglia la spesa sociale e, come l'avevate fatto nel 2004, lo state facendo adesso. Solo durante i Governi Conte abbiamo in parte sbloccato con il decreto cosiddetto Calabria le assunzioni del personale sanitario. La seconda ricetta per accorciare le liste d'attesa è spostare alcune delle prestazioni sul territorio. Ma anche questo evidentemente non l'avete capito se state tagliando 300 case di comunità e 100 ospedali di comunità nel PNRR. Qual è la differenza tra noi e voi? La differenza la fanno i numeri e i fatti. Noi avevamo investito 13 miliardi di euro sulla sanità, più 16 miliardi previsti nel PNRR. Voi, passando dal 7 per cento del PIL in spesa sanitaria al 6,3, avete di fatto bruciato 14 miliardi di euro sulla sanità. Questi sono i dati. Per questo abbiamo depositato una legge che chiede di inserire l'investimento sanitario minimo al 7 per cento, per metterci in linea con gli altri Paesi europei. che i vostri tagli continueranno, non si fermeranno, perché i Governi di austerità questo fanno e, anziché vedere la protezione della salute come un investimento, lo vedono come un costo. Quello che abbiate il coraggio in Europa, dove si discute il Patto di stabilità, di chiedere non lo scorporo delle spese militari, ma quantomeno lo scorporo delle spese sulla prevenzione. La prevenzione, gli *screening* oncologici sono un investimento o sono un costo anche quelli? Oggi leggevo i comunicati usciti dopo le dichiarazioni del Ministro alla Camera, che dice che in realtà in questo DEF c'è anche tutta la programmazione, basta saperla leggere, basta vedere quali sono stati gli investimenti sul lavoro. Forse, però, il Ministro non legge i dati del Ministero del lavoro che dice che il 10 per cento dei nuovi contratti che si stanno stipulando duran un giorno e solo l'uno per cento dei nuovi contratti supera supera l'anno. Quindi qual è il lavoro che state creando? Lavoro povero e lavoro precario. *(Applausi)*. Ha parlato anche di sacrificio. Certo è grande il sacrificio per i cittadini a cui state tagliando la spesa sanitaria, la spesa in istruzione. Certamente non c'è alcun sacrificio per le banche, per gli evasori fiscali a cui continuate a strizzare l'occhiolino, per le squadre di calcio a cui avete dilazionato il pagamento delle tasse. Di investimenti, invece, non c'è assolutamente traccia. Presidente, come al solito, le spese di queste politiche scellerate le pagheranno i cittadini e le pagheranno soprattutto i cittadini più più fragili. Noi siamo dalla loro parte e continueremo invece a sostenere che, soprattutto nei momenti di fragilità, vanno intanto aiutate le persone più fragili, più in difficoltà e a tutti auguro buona festa della Liberazione e viva l'Italia antifascista.

cerchiamo di fare un po' d'ordine. A cosa serve innanzitutto il DEF? Il DEF serve ad avere un quadro delle grandezze macroeconomiche e, sulla base di quello, poi predisporre la legge di bilancio. Ebbene, come va l'economia? Benino. Certo, potrebbe andare meglio, ma va anche meglio del previsto. Guardiamo qualche grandezza. Cominciamo dal PIL, che è la misura dell'economia. per cento quest'anno, ma, al di là del dato, è importante il confronto con i nostri *competitor* europei. Infatti, il modello flessibile dell'Italia va meglio di quelli della Francia e della Germania, strutturalmente motore economico dell'Europa. La Francia ha da tantissimi anni la bilancia commerciale in passivo e questo prima o poi diventa un problema; la Germania vede in crisi il suo modello tradizionale di sviluppo e di economia, che aveva alla base anche un vantaggio competitivo sul costo dell'energia e, quindi, deve rivedere strutturalmente il proprio modello economico;

che è la vera misura di come va l'economia, il vero indicatore e anche il vero e principale obiettivo di politica economica, abbiamo raggiunto livelli *record* di occupazione. Questo è un dato oggettivo. La disoccupazione è calata;

Il debito chiaramente per l'Italia è un problema particolare - come sappiamo - ma è aumentata di molto la quota acquistata dagli italiani e questo è chiaramente un dato di stabilità. Le aste dei BOT vanno particolarmente bene. Abbiamo detto che i tassi d'interesse andranno a scendere.

Insomma, l'economia tiene nonostante i venti di guerra e i molti altri problemi che conosciamo tutti. Questo è di certo merito degli imprenditori, perché l'economia la fanno le imprese e gli imprenditori, ma anche di scelte di politica economica. Vediamo allora quali sono state le principali scelte di politica economica che

La politica è scelta e spesso le scelte giuste sono anche politicamente costose. E questo in teoria, perché - a mio avviso - alla fine la serietà paga sempre; magari nel breve sono politicamente costose, ma nel medio e nel lungo termine la serietà paga. Ad esempio, quando il prezzo della benzina scese sotto i due euro, si è scelto di tagliare subito gli sconti fiscali.

Poi la Lega ha sostenuto altre scelte di politica economica giuste, anche se politicamente costose, anche se - lo ribadisco - solo in teoria, perché alla fine è la serietà che paga, è la credibilità che paga. Così è stata fatta una stretta necessaria e giusta sul reddito di cittadinanza, con è calata la disoccupazione ed è aumentata l'occupazione. Abbiamo il *record* di tasso di occupazione. Quindi, era giusto tagliare il reddito di cittadinanza. Altro esempio: si è data una stretta e siamo alla fine della stagione folle dei *bonus* edilizi. Effetto: scende l'inflazione, ma è logico. Dato il peso del settore costruzioni sull'economia, la stretta sul superbonus inevitabilmente e fortunatamente accelera il calo dell'inflazione. Dell'impatto del superbonus si è già detto molto e non mi dilungo, non ripeto cose stranote. Sottolineo però un aspetto: spesso si parla di *spending review*, spesso si parla di razionalizzazione della miriade degli sconti fiscali (sono 226, a memoria, i crediti fiscali). il credito fiscale altro non è che una mancata entrata e quindi equivale a una spesa. Il credito fiscale è una spesa. Ebbene, quanto vale? Il superbonus - com'è stato detto - vale 220 miliardi; nel periodo, sono 25 miliardi l'anno. È una cifra imponente. La fine del 110 per cento è la madre di tutte le *spending review*: perché se vale 25 miliardi l'anno, chiudere il rubinetto vuol dire non spendere 25 miliardi l'anno. Per non parlare poi dell'effetto che questo ha sul *deficit* e sul debito. Fate solo un esercizio mentale: prendete le tabelline del DEF e rimettete da qui all'eternità il superbonus e aggiungete 25 miliardi in più all'anno. Andiamo a sbattere. Chiudiamo però con una nota positiva sul debito, in particolare, che è la grandezza che più di tutte dobbiamo monitorare. Allora cito Einaudi, visto che parliamo di politica economica sana. Siamo nel Siamo nel 1920 e si parla di debito: cosa dice Einaudi? Lo Stato manterrà fede all'impegno assunto? Molti hanno paura che lo Stato non possa mantenere fede all'impegno assunto di pagare il 5 per cento sui prestiti di guerra sui prestiti di guerra e su quello ora bandito per la pace sociale. L'esperienza del passato dovrebbe in proposito essere ammonitrice. Einaudi allora fa un esempio, perché ricorda che nel 1866 il debito pubblico assorbiva la metà del bilancio

le difficoltà finanziarie odierne, sebbene grandi, non ci devono dunque spaventare. Le supereremo, così come abbiamo vinto quelle maggiori del periodo eroico della formazione dell'Italia. Con questa nota positiva, quindi, auguriamo buon lavoro al ministro Giorgetti, al sottosegretario Freni qui presente, al Governo tutto, con una banale constatazione. Alla fine la serietà paga, sempre.

Il Governo ci racconta cioè come stanno andando le cose, come va l'economia, come vanno i conti pubblici, ma non ci dice nulla su cosa ha intenzione di fare per il futuro; non ci spiega come ha intenzione di impostare, almeno a grandi linee, la prossima manovra di bilancio. Presidente, il Governo politico non ha una politica economica. Questo è quello che emerge da questo DEF. Il Governo che ha l'ambizione di essere un Governo politico e di legislatura si sta comportando come un Governo balneare, come un Governo dimissionario, come un Governo che ha di fronte a sé un orizzonte temporale brevissimo. Signor Presidente, mi lasci un DEF così è una presa in giro nei confronti del Parlamento, una presa in giro nei confronti dell'Italia. Vi è una motivazione ufficiale, che ci è stata ripetuta in tutte le audizioni: c'è il nuovo Patto di stabilità e crescita; mancano alcuni documenti tecnici; non vi era la possibilità di costruire una parte programmatica coerente con le nuove regole. è una scusa che fa acqua da tutte le parti. E fa acqua da tutte le parti perché il Ministero dell'economia ha tutti i numeri, ha tutte le simulazioni ed è perfettamente in grado di costruire un quadro programmatico dell'economia, dei conti pubblici e di quello che sarà l'impatto della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo che sarà aperta - come ha detto il ministro Giorgetti - a partire da giugno. È una scusa che fa acqua da tutte le parti quella con cui il Governo ha motivato il DEF solo tendenziale, perché gran parte dei 27 Paesi dell'Unione presenterà documenti programmatici, anche se c'è il nuovo Patto di stabilità. Signor Presidente, i veri motivi per cui il Governo ha presentato un documento solo tendenziale sono altri. I veri motivi sono che la situazione è difficile e che bisogna tenere coperte le carte, bisogna tirare a campare, bisogna scavallare le elezioni europee e amministrative. È difficile la situazione macroeconomica, perché la crescita del 2024 - come vi avevamo detto già in autunno - è inferiore rispetto alle previsioni della NADEF, con stime che sono state abbassate, ma che sono più ottimiste rispetto a quello che dicono l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, il Fondo monetario internazionale, la Confindustria. Scegliete voi: qualunque previsione è sempre inferiore rispetto a quello che il Governo scrive nel DEF. La situazione macroeconomica è difficile perché la crescita nei prossimi tre anni, nel 2025, 2026 e 2027, è appesa al PNRR, la cui attuazione vale il 90 per cento della crescita tendenziale che avete scritto nel Documento di economia e finanza. Se lo attuiamo - come tutti speriamo è possibile che quegli obiettivi vengano raggiunti; ma, se le cose non vanno, l'Italia si avvierà verso la stagnazione. È difficile la situazione dei conti pubblici, signor Presidente, perché nel 2023 il *deficit* è andato fuori controllo. Era previsto al 5,3 per cento a settembre; è salito al 7,2 nella prima stima; è arrivato al 7,4 per cento con la notifica a Eurostat di pochi giorni fa. Sono 48 miliardi di euro, non bruscolini; 48 miliardi di euro in più rispetto a quello che veniva previsto a settembre. Pesa il superbonus? Certo che sì. A dicembre 2022 il costo era di 69 miliardi: siamo saliti a 100 miliardi a dicembre 2023 e a 122 miliardi a marzo del 2024. andrebbe spiegato che cosa non ha funzionato, perché questo è un Governo che è in carica da diciotto mesi, non da ieri. Ed è un Governo che, a febbraio del 2023, ha bloccato la cessione dei crediti del superbonus, raccontandoci che la situazione era stata riportata sotto controllo. Da allora, mese dopo mese, i costi sono continuamente aumentati e voi vi siete svegliati solo poche settimane fa, quando i buoi erano già usciti dalla stalla. Allora dovete spiegarci e dovete spiegare al Paese che cosa non ha funzionato. Perché avete avuto 50 miliardi di euro di costi in più per il superbonus, quando ci avevate raccontato che avevate riportato sotto controllo la situazione? Male il 2023 e, dal 2024 in avanti, la cattiva notizia è il debito pubblico, che prevedevate in lieve riduzione con la NADEF e invece torna a crescere, fino a sfiorare il 140 per cento secondo i vostri numeri, perché, leggendo l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, i rischi al ribasso, cioè i rischi che il debito cresca ancora di più, sono veramente importanti. Il terzo elemento di difficoltà è il nuovo Patto di stabilità e crescita. Presidente, me lo lasci dire: la destra - Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia - ha dato il meglio di sé. A dicembre la presidente Meloni e il ministro Giorgetti sono venuti in quest'Aula davanti a noi a dire che quello era un accordo soddisfacente, un buon compromesso. È stato detto: l'Italia ha portato a casa molto; certo non è il massimo che avremmo voluto, ma è un accordo soddisfacente. Non siete però riusciti a convincere nemmeno i vostri parlamentari europei che si sono astenuti sul nuovo Patto di stabilità che è stato approvato dal Governo all'Ecofin e al Consiglio europeo. Si sono astenuti perché si sono resi conto che quello non era un accordo così soddisfacente e che l'Italia non aveva portato a casa così tanto. grazie al Patto di stabilità e crescita che avete subito - perché quello è un accordo franco-tedesco - il sentiero è diventato strettissimo. Magari i conti rimarranno allineati a quelli della NADEF e al tendenziale del DEF, come ha auspicato il ministro Giorgetti, però bisognerà trovare lo stesso un sacco di soldi. C'è infatti una tabellina scarna che dice la ciccia di questo Documento di economia e finanza, ed è quello sulle politiche invariate, dove voi scrivete che è necessario trovare 19 miliardi nel 2025, 23 miliardi nel 2026, 25 miliardi nel 2027 - quindi un crescendo solo per confermare quello che il ministro Giorgetti ha chiamato le cambiali - bontà sua - che sono state firmate sulla testa degli italiani quando avete fatto una legge di bilancio che ha finanziato solo per un anno il taglio del cuneo contributivo, solo per un anno la riforma Irpef, solo per un anno persino il taglietto del canone RAI. Quelle cambiali stanno venendo a scadenza e bisogna trovare un sacco di soldi. Non sapete come fare e naturalmente non scrivete come avete intenzione di recuperare quelle risorse. Vanno trovati i soldi per le politiche invariate, ma naturalmente vorrete fare qualcosa di nuovo con la legge di bilancio 2025 e 2027. Guardate che la sanità sta cascando a pezzi e c'è un tema previdenziale; ci sono le politiche per il lavoro, gli investimenti, le politiche industriali. È per questo che tenete le carte coperte: non sapete che pesci pigliare per la prossima manovra di bilancio perché non avete una strategia per rilanciare la crescita che sta tornando allo "zero virgola"; perché non sapete come affrontare i nodi sociali, con la povertà assoluta al massimo storico, con la precarietà e la povertà lavorativa che crescono, con la sanità pubblica che è in crisi profondissima. Non sapete che pesci pigliare perché avete promesso un fisco amico - prendo in prestito una felice espressione di un collega - ma state costruendo il fisco degli amici *(Applausi)*, che mantiene i regimi di favore, che è sempre più indulgente e permissivo verso i soliti noti. Non sapete che pesci pigliare, perché non sapete persino spendere i soldi che avete a disposizione. La presidente Meloni è venuta in quest'Aula a raccontarci che con la revisione del PNRR vengono stanziati oltre 6 miliardi di euro per le imprese (il piano Transizione 5.0). Siamo ad aprile e non ci sono i provvedimenti attuativi; quei soldi sono congelati, sono fermi; sono fermi gli 1,8 miliardi di crediti di imposta per la ZES. Non riuscite a spendere nemmeno i soldi che avete a disposizione per finanziare gli investimenti e la crescita. Allora tenete le carte coperte perché volete nascondere la verità agli italiani: non volete dire quali tasse sarete costretti ad aumentare; quali spese dovrete tagliare con la manovra in autunno. E non lo volete dire adesso, perché tra un mese e mezzo ci sono le elezioni europee. Bisogna andare a prendere i voti e naturalmente non si prendono i voti raccontando la reale condizione del Paese dopo diciotto mesi di Governo Meloni. Questo è il quadro che emerge da un Documento che di fatto è una pagina bianca. È un quadro difficile, È un quadro difficile, ma è un quadro in cui il Governo politico e di legislatura, il Governo che è nato con l'ambizione di cambiare l'Italia, ha deciso che è meglio rimanere in silenzio. Il vostro Governo ha rinunciato a governare e questa non è una buona notizia per l'Italia e per gli italiani. Signor Presidente, mi lasci iniziare questo mio breve intervento con un momento di tristezza, perché vedere colleghi

qualche aggettivo diverso o qualche sinonimo, mi sembra la solita pastetta, che non è ovviamente in nessun modo agganciata alla realtà dei fatti e che vede un mondo completamente diverso, il processo alle intenzioni è la base del ragionamento e il fatto di fare i menagrami sulle spalle e alle spese dell'Italia e degli italiani è la sintesi degli interventi che ho ascoltato fino a qui, da illustri Ne è una prova il dibattito di ieri sul PNRR, basato su una semplice e banale constatazione, secondo cui sarà necessario ragionare con l'Europa, con la rinnovata forza di questo Governo di questo Paese, per chiederle di riconsiderare il termine del 2026, almeno per darci modo e tempo di mettere a terra i lavori avviati e gli investimenti effettuati. Ciò tiene conto di una realtà Paese che oggi "Il Sole 24 Ore" illustra molto bene e molto efficacemente, dicendo che in tre anni la spesa dell'Italia per cento sui fondi della programmazione europea. In tre anni, la programmazione 2021-2027 è stata tirata da questo Paese e dal suo sistema di burocrazia e di regole solo per l'uno per cento. Quindi dire che dobbiamo tentare di affrontare un discorso in sede europea che rimetta in discussione la scadenza del 2026 significa essere italiani, significa essere realisti,

Non esistono i risultati di questo Governo sul versante dell'inflazione, la più bassa di tutti i Paesi europei? Non esistono i risultati di questo Governo sull'incremento di PIL che sta scritto nel DEF, il più alto di tutti i Paesi europei? Mi riferisco all'incremento programmato di PIL rispetto alla programmazione degli degli altri Paesi europei. Non esistono i risultati, perfettamente descritti dal collega Garavaglia, sul tasso di occupazione e sul tasso di disoccupazione, che sfiora il 7 E sì che voi avete avuto risultati straordinariamente più belli, per cui ve ne potete anche vantare. Non esiste lo *spread*, che era lo spauracchio di tutti i Governi fino a ieri e che oggi è in continuo ribasso? Il nostro debito pubblico viene appetito di *rating*. No, tutto questo non esiste. Esistono i processi alle intenzioni, il detto e non detto, che cosa nasconde l'affermazione o la virgola sull'affermazione del Ministro, che cosa è la vostra reale intenzione. Ma, scusate, colleghi, leggete le carte. Capisco che questo DEF è piuttosto corposo, però leggetelo. Vengo ad esempio a parlare della spesa sanitaria. pagina 35 del DEF illustra il totale delle uscite correnti e disegna un percorso che parte nel 2022 con 131 miliardi e arriva al 2027 con 147 miliardi di euro, sfiora i 150 miliardi di euro, cifra da tutti ritenuta come la cifra ideale di dotazione del nostro Fondo sanitario nazionale. Pagina 35 del DEF; leggetele le carte, perché poi non riuscite a commentare i numeri, se non le leggete. Nel quadriennio 2020-2023

secondo nello stesso periodo viene descritto come incrementale del 3,1 per cento, c'è bisogno di essere ingegneri informatici per capire che il rapporto PIL e spesa sanitaria non può che restare su quel livello, perché il PIL incrementa più della spesa sanitaria? *(Applausi)*. Ci volete dire che è un problema del Governo che il PIL incrementa più della spesa sanitaria? Sinceramente non riesco a mettermi nei panni di chi è in grado di descrivere il quadro attuale con tale spregiudicatezza, come la collega Lorenzin, che ha fatto il Ministro in un glorioso periodo di questa Nazione,

senza aver mai vinto le elezioni - questo va detto, a futura memoria - e ci avete consegnato una situazione della sanità che è davanti agli occhi di tutti? La collega Castellone dice che bisogna assumere:

gran parte delle Regioni non ha esaurito la capacità assunzionale prevista dai decreti Covid.

È sotto gli occhi di tutti quello che ci avete lasciato. Ciò che desta in me veramente scalpore è con quale faccia venite a condannarci per le cose che avete fatto voi, dicendoci di fare quello che voi non avete fatto, avete fatto, e perché non facciamo le cose che ci dite che dobbiamo fare. Noi abbiamo vinto le elezioni e voi le avete perse: voi siete stati la malattia e gli italiani hanno scelto il centrodestra perché fosse la medicina;

Mettiamoci allora in linea con i fatti: stiamo lavorando alacremente al rifinanziamento della sanità e stiamo ottenendo risultati importanti sul versante del lavoro, anche con una importante

contrapposizione politica l'interesse nazionale. Lo fate quando parlate dei provvedimenti europei. Noi ieri ci siamo astenuti in Europa proprio perché volevamo di più e quel di più lo otterremo grazie a quell'astensione. Stiamo rifinanziando il Fondo sanitario nazionale, ma dobbiamo ridare fiducia al nostro sistema delle professioni,

basta dare addosso alla salute in questo Paese, perché ci facciamo male tutti, perché, colleghi, sappiate che prima o poi, davanti a quel sistema sanitario, ci finiremo tutti, quindi vi state anche dando la zappa sui piedi. Potete fare le corna, ma così sarà.

Non si tratta di non avere una politica economica, non si tratta di volersi comportare come un Governo balneare o di voler tenere le carte coperte, o addirittura di non sapere che pesci pigliare,

evitare di scrivere sull'acqua un testo programmatico che non avrebbe una sua rispondenza. Non è un caso che il Governo, nell'accettare la proposta di risoluzione della maggioranza, ne abbia accettato l'impegno principale che risponde probabilmente anche a tutte le obiezioni che sono state fatte sino ad oggi, e cioè quello di presentare il quadro programmatico quando quando il piano fiscale strutturale di medio periodo sarà stato elaborato e lo consentirà. Noi possiamo continuare a ragionare con strumenti passati, cercando di costruire questa casa con una cassetta degli attrezzi che non è più attuale,

nefasto della cessione del credito, che è cosa diversa e ulteriore rispetto al solo superbonus. A me piace immaginare la politica economica che un Governo deve portare avanti quotidianamente come una passeggiata in montagna. Chi passeggia in montagna sa bene che ci sono fattori ampiamente prevedibili: si può scegliere l'abbigliamento corretto, magari evitando di andare a passeggiare con le scarpe da città e mettere delle scarpe da montagna, ci si può vestire in modo corretto rispetto alla stagione, ci sono fattori moderatamente ponderabili, si può scegliere un percorso più o meno facile in ragione delle attitudini e ci sono poi dei fattori assolutamente imponderabili. Chi cammina in montagna sa che può avere le scarpe giuste, può avere l'abbigliamento giusto, può camminare sul sentiero corretto per la sua attitudine, ma che una nuvola può arrivare in qualsiasi momento e sbarrare la strada, che può venire un acquazzone in qualsiasi momento. La politica economica è composta da tutti e tre questi elementi. Quando un Governo fa la politica economica di un Paese, amministra fattori prevedibili, fattori irragionevolmente ponderabili e fattori certamente imponderabili.

da nessun Governo nazionale. Di fronte a tali dinamiche (questa è la famosa nuvola che scende a ostruire il percorso), il Governo ha scelto una politica responsabile, che puntasse a preservare il potere d'acquisto dei redditi medio-bassi. Ha scelto questa politica, nonostante in questa nostra metaforica camminata in montagna non solo la strada fosse sbarrata da una nuvola, ma avesse anche cominciato a piovere e questa pioggia - secondo quanto esposto da Banca d'Italia, nell'audizione che ha depositato in Commissione questa mattina - vale l'8 per

219 miliardi di *bonus* edilizi a fronte di 196 miliardi di PNRR. Parliamo di numeri, guardiamoli questi numeri. Il Governo, di fronte a questa nuvola che ha sbarrato il passo, di fronte a questo acquazzone che si è trovato a dover fronteggiare (un acquazzone che, lo ripeto, vale l'8 per cento del PIL) ha scelto coerentemente, insieme all'Europa - così rispondo anche agli amici del Partito Democratico, da cui ho sentito più volte questa accusa, non si può essere europeisti a corrente alternata - di non presentare un quadro programmatico. Tale scelta è stata concordata con la Commissione europea e questo non lo dice Federico Freni, che nulla conta ovviamente, ma la Commissione europea.

dato corso a una politica economica rispecchiata in un DEF certamente responsabile; una politica economica che, per tornare alla nostra passeggiata in montagna, deve consentirci non solo di passeggiare, ma anche di tornare a casa di tornare a casa nonostante la pioggia, nonostante la nuvola, consapevoli di aver scelto - per restare in montagna - le scarpe giuste e consapevoli che non sarà certamente questa nuvola a impedirci di elaborare di elaborare - uscendo di metafora - la politica economica più corretta, che è appunto quella contenuta, quanto al quadro tendenziale, nel DEF che oggi viene votato e, quanto al quadro programmatico, quella che, in ottemperanza alla risoluzione di maggioranza che il Governo ha appena accettato, sarà elaborata non appena il quadro di medio periodo lo consentirà.

il realismo e la serietà. Questo perché, come diceva il senatore Garavaglia, ciò serve per stabilire la credibilità di un Paese, la capacità per lo Stato di mantenere fede agli impegni presi. presi. Noi pensiamo che il DEF presentato oggi dal Governo non sia sbagliato ma sleale, perché è un documento incompleto, dove le cose taciute rispetto al futuro sono enormemente più rilevanti di quelle descritte rispetto al passato e al presente: è una delega in bianco. L'assenza del quadro programmatico, in violazione delle norme di contabilità e finanza pubblica, è stata giustificata sulla base di precedenti del tutto diversi, cioè di scelte di governi dimissionari che non potevano, anzi non dovevano ipotecare le scelte delle politiche economiche dei futuri esecutivi. Non è mai stato fatto dai governi con i pieni poteri, come piace definirli ad autorevoli esponenti di questa maggioranza. Questa assenza è giustificata sulla base dell'incertezza delle regole del nuovo Patto di stabilità, nel momento in cui il DEF era stato predisposto; in realtà, le regole erano chiare e si sarebbero dovute seguire già prima. A proposito del Patto di stabilità, citato da molti colleghi, è vero che tutti i partiti politici italiani, di maggioranza e opposizione, si sono astenuti o hanno votato contro il Patto di stabilità, ma c'è una differenza fondamentale ed è tra chi, per ragioni di politica interna, con una fuga preventiva dalla responsabilità sui conti, per chiari intenti elettorali, si è astenuto, e chi,

la competitività, sostenere le spese in materia di difesa comune e fare gli investimenti necessari per fare davvero la transizione ecologica e quella digitale. allora, è che l'assenza del quadro programmatico nasconde i necessari correttivi sul fronte fiscale e sulla spesa necessaria a finanziarie le promesse che il Governo continua a fare. fare. In vista delle elezioni europee ci dite quanto volete dare, ma dopo le elezioni europee presenterete il conto dei costi e direte agli italiani quanto e dove volete prendere. Il Ministro dell'economia ha dichiarato di voler confermare le misure relative al taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote IRPEF, che ammontano a un costo complessivo di circa 15 miliardi di euro per il 2025, ma non ha specificato con quali fondi, se intende rendere queste due misure strutturali e non ha chiarito quale dovrebbe essere la fonte del finanziamento strutturale. Forse una nuova clausola di salvaguardia IVA? Inoltre, ci sono 5 miliardi di misure previste solo per il 2024 che non sono state citate, tra cui più di un miliardo per il Mezzogiorno relativo alla ZES unica. Lo scenario macroeconomico del DEF risulta essere più ottimistico rispetto alle previsioni di tutte le altre istituzioni: Banca d'Italia, Ufficio parlamentare di bilancio, Istat, Fondo monetario internazionale. Questo scostamento nelle previsioni è probabilmente dovuto al fatto che lo scenario illustrato nel DEF non tiene conto di alcuni fattori di rischio per la crescita. Per rientrare nella metafora del sottosegretario Freni, anche a me piace fare la passeggiata in montagna, io non credo che sia una nuvola a sbarrare la strada, ma credo che sia una tempesta a poter sbarrare la strada. La tempesta alla quale faccio riferimento è la tensione geopolitica per le guerre in Ucraina e Medio Oriente: questa sì che è una tempesta che può sbarrare la strada a chi vuole camminare in montagna. montagna. Rispondo anche al senatore Zaffini. Noi le leggiamo le pagine, tra cui l'articolo 35 del DEF, ma non basta solo citare i dati, bisogna anche comprenderne il senso nel contesto, perché se lei mi cita un aumento della spesa in termini assoluti, ma non la compara al costo dell'inflazione, capirà bene che con quella spesa nel 2024 non ci compra neanche le cose che poteva comprare nel 2019. Ecco perché c'è il tema del rapporto rispetto alla spesa sanitaria e il *deficit*-PIL. Ancora, voglio suggerire al Governo di non usare gli effetti nefasti del superbonus come alibi, ma come sprone per una maggiore e diversa responsabilità, perché il tema del crollo e della voragine nei conti pubblici si può fare sul superbonus per eccesso, ma si può fare anche sulla sanità Noi vi abbiamo chiesto alcune cose, quattro domande semplici all'atto della presentazione del DEF. Vi abbiamo chiesto, in primo luogo: come intendete finanziare le misure fiscali che dite di voler confermare per il 2025? Seconda per quali ragioni le previsioni macroeconomiche del DEF sono notevolmente più ottimistiche delle previsioni di tutti gli altri istituti? Possibile che tutti gli altri istituti si siano sbagliati e solo le vostre previsioni siano quelle giuste? vi abbiamo chiesto cosa intendete fare per triplicare la capacità di spesa della pubblica amministrazione necessaria per garantire la realizzazione degli investimenti del PNRR nei tempi previsti, visto che dovremo spendere ogni anno il triplo di quanto abbiamo speso fino ad oggi. vi abbiamo chiesto se assumete un impegno per prevedere, a partire dalla legge di bilancio 2025, un graduale aumento della spesa sanitaria nel periodo di programmazione per portare il finanziamento a una quota pari all'8

parlare di aumento della spesa, ma concepire e rendere tecnicamente realizzabili azioni concrete per riqualificare la spesa sanitaria; per riqualificare una spesa che consenta di liberare risorse per intervenire in prima battuta e con una certa urgenza sul costo del personale sanitario, sia in termini di aumento del numero dei professionisti, sia per adeguare l'inaccettabile condizione stipendiale. Signor Presidente, queste sono le domande che, come Azione, abbiamo posto a nome dei cittadini al Governo. Queste domande non hanno ottenuto risposta ed è questo il motivo per il quale Azione voterà contro il DEF: perché noi deleghe in bianco a questo Governo non le firmiamo.

che abbiamo dovuto ascoltare nella discussione di oggi, che riflettono la dimensione surreale, *rectius* lunare, in cui le opposizioni paiono trovarsi ogniqualvolta c'è da esaminare un atto fondamentale del Governo, mi induce a voler chiarire alcuni punti fermi, che possiamo rintracciare anche nel Documento di economia e finanza al nostro esame. nostro esame. Ai colleghi delle opposizioni mi corre l'obbligo di ricordare che il DEF non è una legge di bilancio, il DEF non deve trovare i soldi. Il DEF delinea un quadro economico, fa prospettive e tiene conto dell'andamento economico. La fotografia che ci ha fatto il ministro Giorgetti è quindi saggiamente cauta, perché il contesto economico economico che abbiamo di fronte lo conosciamo tutti o, forse, ancora non lo conosciamo affatto ed è quindi complicato fare previsioni. Al momento, però, il contesto è quello di una crisi internazionale con una guerra, con le tensioni in Medio Oriente ed alle nostre porte in Ucraina; è quello in cui la BCE ha aumentato i tassi, quello in cui i costi delle materie prime e del petrolio sono schizzati alle stelle. In questa analisi cauta, giustamente cauta, noi abbiamo avuto comunque un incremento del PIL nazionale, nel 2023, dello 0,9 per cento: addirittura in aumento rispetto alla previsione della NaDEF 2023, che era +0,8 ed addirittura superiore a quella della media dell'area euro, che era +0,4. Questo significa che i consumi delle famiglie, per noi fari nella notte, nel 2023 sono cresciuti ad un ritmo significativo. Ma vi è di più. La previsione tendenziale del tasso di crescita del PIL si attesta, per l'anno 2024, all'uno per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 e allo 0,9, rispettivamente, nei due anni anni successivi. Tale crescita sarà sostenuta, in particolare, dagli investimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie, tenuto conto che l'azione di Governo per il 2024 sta proseguendo in questa direzione. Non lo diciamo noi, ma lo dice l'Istat, come certificano i dati alla mano nel DEF, se solo se aveste avuto la bontà di approfondire meglio le tabelle. Viene allora da domandarsi se questa opposizione sia la stessa del 2020, cioè quella che con i *bonus* edilizi, appunto, ha creato un sistema che ha portato ben 120 miliardi di euro di buco, di debiti fuori bilancio nei conti dello Stato, un numero che continua a crescere ed il cui saldo finale, purtroppo, vediamo salire, come ha detto poc'anzi il sottosegretario Freni, sopra i 210 miliardi. Una cifra *monstre*, addirittura superiore a quella degli investimenti del PNRR. Ce ne vogliamo rendere conto? Colleghi, questi miliardi di euro di debiti fuori bilancio ci ricordiamo bene a cosa sono serviti. Quando si fanno dei crediti d'imposta, le poste vanno messe a bilancio e noi lo abbiamo fatto in tanti provvedimenti. Abbiamo previsto ed appostato, ad esempio, miliardi di euro sul taglio delle bollette, sul credito d'imposta per le aziende e per gli aiuti alle famiglie. Tutte cose che sono scritte nero su bianco, i cui nomi ritornano. Abbiamo previsto una spesa, abbiamo previsto un termine per quella spesa. Quando, invece, si lascia la libertà della trattativa privata, in altri termini si lascia a tutti la possibilità di creare debito per lo Stato

Con quei soldi si è andati ad intervenire - udite udite - sul 2 per cento del patrimonio immobiliare italiano e, tanto per intenderci, noi tutti abbiamo pagato le seconde e le terze case in montagna o al mare ai ricchi, cioè a chi non ne aveva bisogno, con quasi 2.000 euro di debito a testa. Ve lo assicuro, perché anche un mio caro amico, che è miliardario, si è fatto la casa con 700 milioni che gli sono stati regalati dallo Stato. Tanto per essere chiari - lo dico a chi oggi fa finta di avere la memoria corta - con i soldi di tutti, anche di chi abita nelle periferie, abbiamo pagato magari la seconda o la terza casa di chi sta andando comodamente in ZTL, chi può permettersi il *personal shopper* a 300 euro al al mese o magari l'armocromista. Ecco perché non accettiamo lezioni di economia da chi ha sfasciato letteralmente i conti pubblici, perché questo è quello che la sinistra, col portafogli a destra, e i Governi giallorossi ci hanno lasciato: un buco enorme, un debito pubblico pesantemente condizionato nei prossimi anni dai riflessi per la cassa del superbonus, per dirla con le parole del del ministro Giorgetti. Oggi però c'è un Governo che affronta con lucidità i temi macroeconomici in un momento difficile e incerto per il Paese. Questo DEF è un Documento serio che guarda alla realtà del nostro Paese e che permette anche agli operatori del settore di guardare con fiducia al futuro dell'Italia. Questo è un dato importantissimo e lo voglio ricordare, come pure voglio ricordare l'impegno che questo Governo e questa maggioranza si sono assunti, ossia ridurre progressivamente il *deficit* nel prossimo triennio. Dobbiamo e vogliamo lasciarci alle spalle l'impatto devastante dei vari *bonus* edilizi e assistenzialisti che drogano l'economia. Il messaggio che vogliamo dare agli italiani è, al contrario, che la stagione dei *bonus* a pioggia si è chiusa, è finita; che il percorso di riduzione del debito dovrà venire da una crescita economica che la politica di bilancio potrà favorire, ma solo attraverso una ricomposizione della spesa pubblica e dei prelievi fiscali, non con altro e soprattutto non con nuovo debito. Questo è quello che ci dice questo DEF, e lo dice in modo forte e chiaro. Colleghi, statene certi, mentre voi starete ancora elaborando il lutto per il caro estinto, quel famoso "tutto gratis", noi staremo costruendo una nuova politica fiscale, tagliando il cuneo e riducendo la pressione fiscale sui cittadini e le imprese. Staremo costruendo, ad esempio, nuove politiche per la sanità pubblica, per la quale in termini assoluti nel DEF si prevede una spesa sanitaria di oltre 138,7 miliardi, cioè 7,6 miliardi in più rispetto al 2023. In altre parole, avremo il 6,4 per cento del PIL investito in sanità: un valore mai così alto. A differenza della vostra narrazione, questi sono numeri, *ergo* fatti. Venendo invece al capitolo della produzione industriale e al mercato del lavoro, nel DEF leggiamo indicazioni molto favorevoli che derivano dal clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Non a caso, le politiche di questo Governo di centrodestra si sono concentrate nel dare un sostegno ai redditi dei lavoratori prevalentemente, ma anche riducendo la pressione contributiva, e questo ha consentito alle famiglie di recuperare il loro potere di acquisto dopo la fiammata inflazionistica. Questo avevamo promesso agli italiani, ossia dare solide certezze alle famiglie e una solida attuazione patrimoniale, perché i cittadini ci chiedono certezze, normalità, misure strutturali, programmatiche e di legislatura. Siamo orgogliosi per la fiducia che infatti continuano a darci

la discontinuità e, invece che mettere le mani nelle tasche dei cittadini, nella scia tracciata a suo tempo dal presidente Berlusconi fin dal 1994 ha il coraggio di impiegare le maggiori risorse in via prioritaria nel tagliare le tasse e dare sostegno al reddito e alla natalità. Quindi credo che il 1° maggio dovremmo tutti festeggiare per quello che sta facendo questo Governo per le fasce più deboli e per i lavoratori onesti. Rinnoviamo quindi la nostra piena fiducia e ringraziamo il presidente Meloni, il ministro Giorgetti, il Sottosegretario qui presente e il Governo tutto per quello che stiamo facendo tutti insieme per questo nostro amato, ma bistrattato Paese.

Signor Presidente, Governo, colleghi e colleghe, partirei con la metafora del sottosegretario Freni, perché noi che proveniamo dalla montagna - il senatore Spagnolli anche dalle alte quote - sappiamo che nessuna nuvola ferma chi sa veramente andare in montagna. Molto spesso chi sa andare in montagna va anche nelle bufere di neve, soprattutto se deve fare soccorso alpino nei confronti di quelli che sono sostanzialmente impreparati ad andare in montagna. Una valanga può bloccare il cammino, non certo una nuvoletta; dobbiamo, in ogni caso, saper tornare a casa anche dalla bufera e dalle difficoltà. Chi fa la guida sa bene che una spedizione deve saper mantenere la rotta e, soprattutto, conoscere la meta che si intende raggiungere. Poi credo che ci sia stato un *lapsus* della collega Biancofiore: doveva essere veramente una bella casa, se sono stati spesi 700 milioni di euro per ristrutturarla. Presidente, sinceramente, venendo invece all'argomento di oggi, non ci convince l'argomentazione delle nuove regole europee rispetto alla mancata presentazione del quadro programmatico. Innanzitutto perché le linee generali del nuovo Patto di stabilità sono già state fissate e i Paesi, come l'Italia, in procedura di *deficit* eccessivo saranno vincolati a ridurre il *deficit* strutturale di mezzo punto di PIL l'anno. Poi è chiaro che in autunno avremo un quadro più definito delle regole e del complessivo contesto economico, ma per quello ci sarà sicuramente la Nota di aggiornamento. Ne consegue che la mancata presentazione del quadro programmatico rende lecite le congetture sull'intento del Governo di superare lo scoglio elettorale prima di dire agli italiani come stanno le cose, ossia che, siccome il Governo non può venir meno agli impegni di riduzione del debito, dovrà necessariamente tagliare servizi e prestazioni o aumentare le tasse. I membri del Governo fanno professione di ottimismo, dicendo che il taglio del cuneo fiscale, le nuove aliquote IRPEF e tutte le altre misure introdotte con l'ultima legge di bilancio verranno confermate. Allora va da sé che l'agnello sacrificale sarà la sanità, saranno saranno i servizi socio-assistenziali e saranno soprattutto le pensioni, con la cancellazione degli scivoli pensionistici, già fortemente ristretti con l'ultima legge di bilancio. In questo ha ragione il ministro Giorgetti nel dire che i bonus edilizi hanno creato una voragine. Ma cosa ha fatto in concreto il Governo per bloccare questo dissanguamento delle finanze pubbliche? cento dei 220 miliardi sono maturati nel 2023, quando cioè questo Governo era già in carica da diversi mesi. E ancora, perché non si è avviato un negoziato in Europa per diluire gli oneri dei bonus su scadenze più lunghe, al fine di ridurre il rapporto debito-PIL già dal 2024, tagliare la spesa sugli interessi e spingere la crescita? In realtà, se si vuole fare un intervento serio sui *bonus* edilizi, non rimane altra strada che quella di semplificare le norme e le tipologie di *bonus*, riconducendole ad unità e definendo normativamente un profilo legislativo, amministrativo e fiscale che sia stabile per almeno dieci anni. Forse sarebbe meglio che rimanesse stabile anche per venti, perché è impossibile pensare ad un risanamento del patrimonio edilizio, finalizzato a contenere i costi di gestione per le famiglie e le persone, senza una stabilità delle norme e senza ovviamente dissanguare i conti pubblici. I *bonus* edilizi quindi non possono diventare un alibi, perché le risorse si possono trovare; serve solo la volontà politica di contrastare l'evasione fiscale, la quale non si combatte solo attraverso l'Agenzia delle entrate, ma anche evitando messaggi su condoni e sanatorie, che generano l'idea di un generale allentamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Ma quel che più ci preoccupa, Presidente, è che nelle scelte di indirizzo economico mancano del tutto le politiche espansive, cioè quelle che danno impulso a una crescita che, come vediamo, è tornata ai livelli pre-pandemia, a quando l'Italia era sempre al di sotto della media europea. L'economia è dentro una trasformazione storica, con l'intelligenza artificiale, i nuovi assetti geopolitici e la trasformazione di interi comparti produttivi nell'ottica della sostenibilità ambientale. Dove sono le misure e gli strumenti per aiutare il nostro sistema produttivo a essere competitivo rispetto a queste grandi sfide? Dove sono l'impegno per riformare lo Stato sociale, con la trasformazione del mercato del lavoro e la richiesta di nuove competenze, la riqualificazione dei vecchi lavoratori e la messa a terra di ammortizzatori sociali, per reggere l'onda d'urto di cambiamenti così profondi? Dov'è il lavoro per liberalizzare quei settori economici ancora viziati dalla presenza di interessi corporativi e di rendite di posizione che ne strozzano lo sviluppo?

Dovremmo parlare più frequentemente della minaccia che per le nostre esportazioni costituisce quanto sta accadendo nel Mar Rosso e della perdita di importanza dei porti italiani a favore di quelli del Nord Europa, dell'aumento dei costi e delle ricadute inflattive. Dovremmo prestare più attenzione al tema delle materie prime critiche, sostenendo il lavoro di chi ne è alla ricerca e l'attività di riciclo e riutilizzo di quelle in disuso, con una forte economia circolare. Dovremmo cioè affrontare tutto quello che oggi è a monte e che costituisce il principale ostacolo alla nostra futura crescita e del modo con cui tutto questo possa tramutarsi in atti concreti, in misure già con la prossima legge di bilancio. Qui invece si sceglie di non farlo e si rimanda la questione all'autunno. Se c'è un messaggio positivo, è soltanto nell'impegno a ridurre il debito. Ci preoccupa e molto la strada che già si intravede, che non è quella coraggiosa della crescita e della lotta all'evasione fiscale, ma quella bassa bassa e poco utile dei tagli e delle nuove tasse. Se andassimo a vedere nella storia economica dell'Italia il periodo di maggior sviluppo del Paese, vedremmo che si tratta di quello in cui c'erano un basso rapporto PIL e debito pubblico e soprattutto un grande risparmio privato. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario al Documento di economia e finanza. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, «Questa sera si recita a soggetto» il titolo di una famosa opera teatrale scritta da Luigi Pirandello, andata in scena per la prima volta in questa città nel 1930. Pensi un po' all'ironia della storia, signor sottosegretario Freni: la compagnia che mise in scena per la prima volta quest'opera era di proprietà di un impresario che si chiamava Guido Salvini. Cosa diceva Cosa diceva quest'opera teatrale? Indagava sull'autoritarismo del regista, speculava, approfondiva e interrogava il rapporto degli attori con il pubblico e soprattutto articolava una messa in scena senza un copione predeterminato, appunto a soggetto, inventando. Ebbene, se volessimo traslare dal genio di Pirandello alla nostra realtà quotidiana, potremmo dire che in qualche misura si indaga, se non proprio sull'autoritarismo del regista di questo Governo, quantomeno sulla sua postura volitiva, sulla sua attività determinata, sulla postura presidenziale della Presidente del Consiglio, che non manca mai di rivendicare, anche come momento di cesura rispetto al passato, la capacità sua e di questo Governo di assumere finalmente decisioni precise, nette e chiare, nell'interesse supremo della Nazione, naturalmente. Potremmo anche parlare del rapporto degli attori delle forze politiche con il pubblico, in una politica oramai ansiogena, sempre alla costante e continua ricerca di una permanente legittimazione in ogni suo passaggio, forse perché intimamente convinta di non essere all'altezza della curva storica chiamata ad attraversare e vivere. Lo stiamo vedendo anche nel modo in cui verranno composte le liste elettorali delle prossime uno sforzo di ricerca legittimante perché evidentemente si sente il bisogno di trovare qualcosa che non sia dentro di sé. Ma soprattutto, visto che parliamo di economia, è una messa in scena occasionale: non imparando a memoria le battute, gli autori le creano da sé e inventano, perché basterebbe leggere l'*incipit* della relazione che voi avete consegnato a questo Parlamento per chiuderla qui la discussione. scrive: «Gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo entro il prossimo 20 settembre». La potremmo anche chiudere qui questa discussione, siete venuti a dirci nulla, forse perché nulla pensate.

Ci avete detto che la crescita il prossimo anno sarà l'1,2 per cento. Poi vi siete dimenticati di prendere il foglio del come, ma in questo forse Crozza vi potrà correre in aiuto. Ci avete detto che il *deficit* si ridurrà dal 2025, anche qui dimenticandovi di spiegare come questo sia possibile e poi avete detto che il rapporto *deficit*-PIL insidiato quest'anno dalla vicenda del superbonus, tornerà in condizioni ordinarie a seguire dal successivo anno rispetto al 2025. Insomma, la fantasia al potere. Intanto, la realtà incede, arriva, è dietro l'angolo e voi la conoscete bene. La realtà drammatica è che l'anno prossimo questo Paese sfonderà il tetto psicologico dei 3.000 miliardi di debito pubblico, perché non avete fatto nulla per fermare questa dinamica. La realtà è che dall'anno prossimo serviranno 20 miliardi per prolungare le misure temporanee che avete introdotto all'interno delle misure approvate *una tantum* all'interno di questo Parlamento. La realtà è che è dietro l'angolo la procedura di *deficit* eccessivo che scatterà per l'Italia dopo le elezioni. Voi avete bisogno di scavallare le elezioni europee e per questo vi siete presentati qui con un foglio bianco e con un racconto inesistente. *(Applausi)*. Il principale epigono di questo racconto è stato un passante, perché se qualcuno, forse scendendo da quelle montagne a cui faceva riferimento nella sua irenica descrizione il sottosegretario Freni, ascoltasse il ministro Giorgetti, potrebbe definire il Ministro dell'economia e delle finanze nel nostro Paese un passante.

ma è stato nel Governo prima come Sottosegretario del Governo Conte 1 - quello del reddito di cittadinanza, sottosegretario Freni, non so se questo le dice qualcosa e poi come Ministro dello sviluppo economico del Gabinetto Draghi. Insomma, il ministro Giorgetti, che adesso viene qui e ci racconta che la colpa è tutta di quelli che sono venuti prima, dovrebbe un po' fare pace con sé stesso: o era un *avatar*, oppure c'è qualcosa che non funziona più in questa dissociazione di chi ci viene a spiegare che la colpa è sempre di quelli di prima, che casualmente, contingentemente sono quelli di adesso, dicendoci molto del livello di deresponsabilizzazione della cifra di questa politica e di questa classe dirigente. Nel 2023 Giorgetti il passante era Ministro dell'economia: è venuto in quest'Aula e ci ha detto che, per gli effetti deprecabili e deprecati del superbonus, eccetera, (superbonus (superbonus prorogato da quel Governo di cui lui faceva parte), si sarebbe dovuto mettere mano alle casse per 13 miliardi aggiuntivi. Questo nel 2023. Quest'anno è venuto e ci ha detto che nel 2023 si è dovuto mettere mani alle casse per 64 miliardi. Scusate, ma visto che c'eravate solo voi nel 2023, chi li ha sbagliati questi conti e come mai adesso ci venite a raccontare questa storia? *(Applausi)*. La verità è che, per la vostra responsabilità, 18 miliardi di tasse. Se lo vogliamo dire in modo un po' più comprensibile, 100 euro al mese per ogni famiglia, perché è evidente che l'incrocio di tutti questi aspetti e il fatto che voi non ci state dicendo come interverrete produrrà un'operazione di questo genere, cioè un aumento di tasse, con buona pace di tutte le chiacchiere che avete fatto e che farete nelle prossime settimane. Anche a Giorgetti il passante ci è venuto a dire in Parlamento che il debito costa, che il debito non buono non va bene, perché lascia un'eredità alle future generazioni. Se ci fosse qui il presidente Monti avrebbe un sussulto davanti a quest'affermazione del ministro Giorgetti. Poi i senatori del suo partito ieri in quest'Aula sono venuti a spiegare che non esiste il debito, perché emettere debito è rimettere in circolo l'economia, anzi fa bene fare debito.

ci trasmette esattamente quello che Kierkegaard descriveva con una bellissima frase che è la descrizione icastica di questo Governo: la nave è ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma il menu del giorno. Per questo voteremo contro

nella mia dichiarazione di voto sarò ancora più fermo nella mia convinzione che il fatto di non aver presentato dei numeri del DEF è una scelta non solo grave e irresponsabile, ma che di fatto vuol nascondere agli italiani prima delle elezioni (quindi è una scelta politica elettorale)

di aver fatto un accordo con l'Europa, in sostanza quell'accordo che ieri i Gruppi parlamentari

con un Documento vuoto, come stanno i fatti. Quindi, è inutile spiegare e leggere i dati, quelli li leggiamo tutti. Vorrei rispondere a qualcuno che ci ha spiegato prima che non capiamo bene come funzionano le cose, compreso il superbonus, perché non mi risulta che molti di voi stessero all'opposizione. Certo, la forza di maggioranza oggi era all'opposizione, ma molti altri stavano al Governo

anzi, tutte le volte peggiorando la situazione, perché tutti gli interventi fatti in termini parziali hanno fatto sì che si accelerasse la

hanno contribuito ad alzare il PIL di questo Paese e a produrre ricchezza. Oggi ci presentate una proposta che è molto al di sotto, perché l'unico momento di crescita è avvenuto

insisto su questo dato. È ovvio che siamo in una situazione in cui rischiamo di perseguire un ragionamento "lacrime e sangue" sulla pelle dei lavoratori, perché anche qui svendete il fatto di intervenire sulle

mentre vorrei sottolineare che il 1° maggio lo festeggerò mobilitandomi e partecipando a manifestazioni insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, che sono in

12 milioni di lavoratori. Io manifesterò con quei lavoratori per chiedere il rinnovo contrattuale. Vorrei capire cosa facciamo tutti insieme, il Governo in particolare, per favorire il rinnovo di quei contratti, in particolare in modo equo, che non si rinnovano per la difficoltà della situazione. Cos'è che si favorisce in quell'indirizzo? Nello stesso tempo, la cosa che vorrei sottolineare dove si vanno a prendere i soldi? Sostengo un altro elemento che ho già ripetuto più volte. Il problema è che bisognerebbe parlare, ad esempio, di chi paga maggiormente in questa situazione. Dovrebbe pagare - secondo

Questo è un dato sancito dalla Costituzione antifascista, per cui domani molti si mobiliteranno nel Paese. Occorre dare una risposta in questi termini, rispettando in sostanza

E se smettono di contribuire coloro che hanno un reddito fisso, questo sarà un problema grave per tutti. Quindi, evitiamo di continuare a discutere

Signor Presidente, il Documento di economia e finanza ci appare molto responsabile, con numeri veri. Prende atto perfino del fatto che il 2023 dovrà registrare un *deficit* di bilancio del 7,4 per cento invece del 5,3. Ciò anche a causa della politica del "gratuitamente", che ha portato a costi notevoli per alcune misure che, se potevano apparire virtuose all'inizio, poi, nella loro prosecuzione, si sono accompagnate a tante violazioni e a tante truffe. Oggi, i due punti di percentuale del *deficit* sono dovuti al superbonus. Il Governo Meloni ha dovuto quindi avviare una politica responsabile, già dai primi suoi passi, e con diversi decreti economici ha cercato di rimettere la situazione sulla giusta carreggiata. L'utilizzo diligente ed efficiente della spesa pubblica deve ancora, però, fare i conti con la condotta disinvolta degli anni passati: passati: quando il Patto di stabilità e crescita europea era sospeso e, un po' per le emergenze in corso e un po' per le scelte sbagliate, che pure ci sono state, la situazione si è in qualche maniera compromessa. Questo Esecutivo e anche il Parlamento con il suo lavoro emendativo hanno cercato, in questo anno e mezzo circa, di mettere in campo misure concrete per il rilancio dell'economia: misure per la famiglia, misure per l'occupazione, misure per le imprese. La decontribuzione, che dovrà proseguire anche nel prossimo anno con dieci miliardi, è una delle misure fondamentali. Anche sulla spesa sanitaria si fanno molte polemiche, ma la realtà è che questa spesa è passata, dai 131 miliardi nel 2023, ai 138,7 miliardi nel 2024, con programmazione di incremento ulteriore negli anni successivi, arrivando quasi a 148 miliardi nel 2027. Quindi, un impegno concreto per la salute. Anche quelli che fanno le valutazioni in riferimento al prodotto interno lordo,

la spesa è significativa e importante. Poi, la sanità è un campo nel quale si deve continuare a lavorare col territorio e con le Regioni. Quindi, c'è chi ha fatto della politica del "gratuitamente" e della irresponsabilità la propria scelta e chi invece cerca di dare un sostegno all'economia reale e all'occupazione. Abbiamo anche affrontato il tema del PNRR. In questi giorni siamo tornati con altri provvedimenti. Le rate sono state pagate, il Piano è stato riscritto molto più puntualmente, con maggiori risorse: oltre 194 miliardi. C'è stata l'azione di un Governo che è venuto sempre in Parlamento a rispondere puntualmente, ad accompagnare i provvedimenti, ad esaurire le richieste dei parlamentari. I piani precedenti, dei Governi Conte e Draghi, erano stati semplicemente respinti al mittente per inattendibilità: questa è la realtà della cronaca recente. *(Applausi)*. Allora, colleghi, è chiaro che ci sono delle incognite. Anche per quanto riguarda la polemica sul Patto di stabilità, trovo assolutamente logico che, di fronte a una nuova stagione che si apre in Europa (si voterà l'8 e il 9 giugno, ci sarà una nuova Commissione europea e ci sono dei temi aperti), la revisione del Patto forse è più giusto che la debbano affrontare la prossima Commissione e il prossimo Parlamento europeo. Riteniamo altresì che alcune direttive sulla transizione ecologica, sulla casa, sull'automobile, sui temi dell'agricoltura debbano essere riesaminate. Forza Italia farà il suo dovere, perché sta nel PPE, che sarà il gruppo politico più numeroso e più importante anche nella prossima legislatura e che potrà indicare, con il rispetto di tutti i grandi tecnici italiani ed europei di ogni Paese, il Presidente della Commissione europea, nell'alveo della politica e del PPE. Quindi è ovvio che in Europa, a fine legislatura, a fine mandato dalla Commissione, anche le vicende di queste ore hanno creato qualche discussione, si guardi più al futuro. In conclusione, signor Presidente, noi vogliamo ricordare, al di là delle proposte di risoluzioni, del DEF e della provvisorietà di esami che saranno poi ripresi con la legge di stabilità con situazioni più definite, che noi questi mesi e in questi anni registriamo: 700 miliardi di titoli di Stato in mani italiane; un *record* storico del BTP Valore; abbiamo lo *spread* a 134 punti, ossia molto al di sotto di epoche passate; è aumentato il tasso di fiducia dei consumatori; ci sono stati 523.000 posti di lavoro in più, quindi non l'assistenzialismo fallito del reddito di cittadinanza ma la creazione di posti di lavoro. Il lavoro è la prima emergenza, è la prima necessità di un Paese; non l'elemosina, la precarietà, l'inganno e lo sperpero, ma la creazione di lavoro,

le bandiere della Palestina e di Hamas si ricordino che i fondamentalisti mettono in crisi i commerci internazionali. Quei droni degli Houthi che attaccano navi che portano merci stanno avvelenando l'economia mondiale *(Applausi)*, non soltanto le vite delle persone. La libertà dei commerci è la premessa per la ricchezza delle Nazioni: questa è una concezione liberale, altro che i droni con le bombe dei fondamentalisti, che sono tutti collegati dall'Iran, agli Houthi dello Yemen e ad Hamas. Credo che domani qualcuno si debba ricordare che si celebra la festa della liberazione dell'Italia e dell'Europa dal nazifascismo, non la festa di Hamas *(Applausi)*, come qualcuno sembra di avere deciso in qualche università. Noi onoriamo quella festa e quella scadenza, e non prendiamo lezioni, perché sono altri che la stanno trasformando in un'altra cosa, con punte di antisemitismo che anche oggi nel servizio pubblico radiotelevisivo sono emerse. Voglio solidarizzare anche qui

della storia, perché la pace l'hanno realizzata uomini come Berlusconi che parlavano con i cattivi del pianeta *(Applausi)*, con i soggetti pericolosi, con i Gheddafi o con i Putin. Parlare di pace con i buoni è facile; portare al tavolo della pace i riottosi, quello è pacifismo, non aggredire i poliziotti in nome del Anche da questo punto di vista concludo l'intervento dicendo che oggi ringrazio il ministro Zangrillo e i Ministri che con lui in queste ore, precisamente alle 16, siederanno al Ministero della funzione pubblica con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, per aprire le trattative per il nuovo contratto per le Forze di polizia grazie ai soldi che questo Governo ha messo nella legge di stabilità dello scorso anno (più di 1 miliardo) e che noi abbiamo anche contribuito ad integrare in Senato. Quel contratto i Governi precedenti non lo hanno rinnovato *(Applausi)*, perché forse stanno dalla parte di chi aggredisce

apprezzabile e crea occupazione. Ci auguriamo inoltre che con l'aiuto di un'Europa che sia madre dei suoi popoli e non matrigna, questa politica possa crescere a ritmi diversi. E ci auguriamo anche, se qualcuno smetterà di seminare odio e guerre nel pianeta, che si possa festeggiare davvero la liberazione non solo del passato, che ricordiamo, ma quella di oggi da guerre, conflitti e dal bisogno. La politica economica serve infatti a creare lavoro, occupazione, sviluppo e benessere. Per questo, voteremo convintamente a favore.

È iscritto a parlare il senatore Monti. del Governo nello scrivere questo secondo DEF. Oggi discutiamo infatti un Documento di economia e finanza in bianco, carente di informazioni, vuoto di contenuti, reticente nei suoi aspetti programmatici e nei suoi aspetti essenziali. Si rinvia tutto a settembre. La verità è che il Governo non ha avuto il coraggio, prima delle elezioni europee, di dire agli italiani che arriveranno tagli e tasse, per la disastrosa politica austeritaria che in questi diciotto mesi il Governo ha attuato. Si sta così occultando l'incapacità del Governo a programmare il futuro del Paese questo DEF lo dimostra tutto. Non era mai successo, Presidente, che un Governo non dimissionario rinunciasse a programmare il futuro del Paese; eppure negli ultimi anni sono state tante le crisi che sono state affrontate. Un grazie va anche rivolto al ministro Giorgetti, perché finalmente nelle audizioni ha detto qual è la politica economica del Governo, qual è la linea economica che il Governo intende seguire:

il neoliberismo, con la sua politica restrittiva, con una scarsa crescita, con il processo di privatizzazione che questo Governo ha già annunciato, così ambizioso, di alcuni *asset* strategici, con la precarizzazione del lavoro, con il lavoro povero, con uno Stato sociale ridotto ai minimi termini e con uno Stato che non c'è più.

L'atteggiamento che pervade l'intero DEF è proprio quello dello studente impreparato, che di fronte alla cattedra dell'arcigno professore prende tempo, racconta che è tutto a posto e che mostrerà il quaderno con tutti i compiti fatti a settembre.

circa 20 miliardi solo per confermare le misure adottate nell'ultima legge di bilancio, tra cui il cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote fiscali, a cui si aggiungono però anche 13-14 miliardi per il rientro del *deficit*. Poi il Governo dovrà anche spiegare al Paese che ha già programmato una riduzione forte della spesa primaria 2024-2027 di circa 70 miliardi di euro, perché la spesa primaria passerà dal 47,2 per cento al 44 per cento del PIL (oltre tre punti percentuali). dello scenario prefigurato nel DEF, noi ci chiediamo come farà il Governo a finanziare la riforma della non autosufficienza, i livelli essenziali nel sociale e nella sanità, così come l'autonomia finanziaria, la riforma fiscale, la *flat tax*, il superamento della legge Fornero e l'abolizione delle accise sulla benzina. Tutte ipotesi e tutte promesse al vento. Anche in questo caso il Governo Meloni ricorre ad un espediente: è sempre colpa di qualcun altro. In questo caso nelle audizioni abbiamo ascoltato il ministro Giorgetti parlare della congiuntura internazionale, delle nuove regole del Patto di stabilità e soprattutto del famigerato superbonus. Io parto da quest'ultimo tema, il male di tutti i mali, bandiera del MoVimento 5 Stelle che noi difendiamo, anche se l'avremmo gestito diversamente da come è stato fatto,

però in quei sei mesi di Governo Conte II noi eravamo in quei parametri prefissati. È stato prorogato nel corso del Governo Draghi, con il voto dell'attuale maggioranza, e poi anche modificato, nel febbraio 2023, dal Governo che non l'ha bloccato, non l'ha cancellato, ma ha posto delle restrizioni che hanno prodotto la corsa all'accaparramento. Questo è quello che è accaduto. Avete sbagliato inoltre le previsioni sul superbonus nel DEF 2023 perché avete previsto una spesa sul superbonus di circa 17 miliardi, che poi è schizzata per la mancanza del monitoraggio concomitante, che noi avevamo già proposto nel corso del Governo Draghi, ponendo un tetto, andando a revisionare le percentuali e anche i destinatari; proposte che il MoVimento 5 Stelle ha avanzato già nella scorsa legislatura, ma che non avete accolto. avete parlato di un buco di bilancio di 200 miliardi; buco che non c'è sia perché nessuna delle autorità istituzionali lo ha accertato, sia perché i mercati finanziari sono tranquilli; tant'è vero che lo *spread* è ai minimi storici. quindi di illazioni. Però, Presidente, con riferimento a questo tema, parlate solo della parte del costo, perché siete ossessionati dal costo debito. Vorrei però ricordarvi che, a fronte di quel costo e del segno dare, c'è anche un segno avere che dimenticate sempre. Il segno avere della crescita *record* del PIL in tre anni, che supera il 13 per cento, delle entrate fiscali aumentate di 140 miliardi, dei posti di lavoro incrementati di oltre 900.000 unità, del debito pubblico che si è ridotto di oltre 17 punti grazie alla crescita *record*. Secondo tema: il Patto di stabilità. Con riferimento all'impatto di tale misura sul DEF, il Governo ricorre alla scusa sempre equiparabile dello studente impreparato che dice che è inutile studiare adesso quando a settembre cambieranno i libri di testo. Tradotto: inutile fare adesso programmazione economico-finanziaria quando a settembre cambieranno le regole sul rientro del debito e del *deficit*. Il Patto di stabilità si preannuncia un patto dell'austerità; questo è quello che voi avete supinamente accettato e votato.

È stato però il miglior accordo possibile per le oligarchie finanziarie che stanno dietro ai vostri partiti. Questa è la santa verità. Si tratta scellerato di lacrime e sangue che costerà agli italiani oltre 13 miliardi l'anno. In ultimo, Presidente, con riferimento al *deficit* del 7,4 per cento, un vero primato per il Governo Meloni in Europa, questo è il risultato che ha portato l'Italia a essere tra i primi in Europa. Tre sono i motivi essenziali di quel 7,4 per cento che neanche avete avuto la capacità di prevedere: l'azzeramento della crescita (zero virgola), l'effetto panico per il decreto sul superbonus, che ha fatto correre all'accaparramento, e poi l'artificio contabile del ministro Giorgetti, che ha spinto Istat

l'unica speranza che abbiamo è il PNRR, ma anche quello state distruggendo. Ormai non è più un piano di ripresa e resilienza, ma sta diventando sempre di più un piano di ritardi e rinvii di spesa realizzata sulle somme ricevute, pari a circa 40 miliardi. Sapete però quant'è la reale spesa realmente in questi diciotto mesi al Governo Meloni? Solo 8 miliardi, perché la restante parte l'abbiamo realizzata grazie al superbonus e Transizione 4.0. Transizione 4.0. Vi sono altri aspetti: innanzi tutto, manca nel DEF la politica industriale, nel momento in cui qui assistiamo ogni giorno alla desertificazione industriale del Paese, ma soprattutto del Mezzogiorno. Lo stabilimento ex Ilva è l'esempio emblematico del fallimento della politica industriale

qualcuno dimentica che abbiamo i salari più bassi d'Europa, che sono fermi da oltre trent'anni e che abbiamo la questione dei salari poveri, quindi una vera e propria emergenza. Attenzione, però: c'è il tema dell'inflazione, ecco perché i salari non possono aumentare. Forse dimenticate che quella di oggi è un'inflazione da costi di approvvigionamento, ma soprattutto da profitti che non avete avuto il coraggio di tassare.

e, quindi, si è autorimandato a settembre. In attesa di affrontare l'arcigno professore, oggi però è meritevole di una sonora bocciatura da parte del Paese.

Signor Presidente, come sempre, avere i colleghi del Movimento 5 Stelle che fanno il loro intervento prima del mio mi fa dimenticare quello che volevo dire. Ho visto Ho visto così, giusto per creatività, che abbiamo sdoganato il termine "austeritario", che sul dizionario non c'è: sarà un austero autoritario, suppongo, o una roba del genere. poi scoperto che son diventati tutti antieuropeisti, dopo essere stati decisivi per votare la von der Leyen: va bene, basta saperlo.

non bisogna buttar via tutto, perché almeno ci dà l'opportunità di passare qualche minuto a parlare di economia. Se ve ne rendete conto, da un po' di anni a questa parte - direi che veleggiamo verso i qui di economia pratica si parla poco. Il Parlamento è sempre più portato a passare del gran tempo in minuzie, le grandi manovre, quello per cui in teoria un Governo, un Parlamento, un periodo possono essere ricordati nella storia, ahimè non si fanno. Cerchiamo di capire velocemente perché, così almeno siamo tutti un po' più consapevoli.

Paesi che dipendono da materie prime - sono così "fortunati" da avere petrolio, gas o altre risorse - e dipendono dal prezzo delle materie prime: se il gas o il petrolio scendono di prezzo, quei Paesi spesso e volentieri si trovano in difficoltà; mentre in periodi in cui internazionalmente il prezzo di quella materia prima va molto bene, ecco che il Paese ha una un periodo di prosperità, indipendentemente da cosa faccia il Governo. E allora cosa può fare il Governo di uno di quei Paesi? Può, ad esempio, cercare di ridurre la dipendenza dalle materie prime e fare una sua politica industriale, che è esattamente ciò che stiamo mettendo su un piatto d'argento alla Russia con le sanzioni. Quello era un Paese che aveva soltanto le materie prime di importazione e le sanzioni l'hanno costretta a fare la cosa giusta, vale a dire a farsi in casa i prodotti e non prenderli da noi.

quel caso la valuta scende e allora, poiché il Paese in quel momento è in difficoltà, i prodotti diventano più convenienti e il Paese un po' si risolleva. È quello che succedeva in Italia prima dell'euro. Altrimenti, quando l'economia di un Paese va molto bene - come succedeva, per esempio, in certi momenti alla Germania - la sua moneta sale, i suoi prodotti diventano troppo costosi, ed ecco che la crescita diventa un po' più tranquilla. In questo momento, non possiamo avere la leva del cambio e allora cosa succede? Bisogna guardare il saldo commerciale e vedere se esportiamo di più di quello che importiamo o meno. In questo caso, noi siamo messi bene: il nostro saldo commerciale è positivo. Altri Paesi all'interno dell'Unione europea non sono messi bene, come la Francia, che in questo momento importa molto di più di quello che esporta, e ci sono Paesi che continuano a esportare tantissimo, come per esempio la Germania.

- che qui andrebbero fatte, ma in questo caso neanche possiamo fare quelle, tranne nei momenti in cui qualcosa scappa fra le righe. fra le righe. Arriviamo così alla questione del superbonus, che è stata forse la più dibattuta. Quando qualcosa scappa fra le righe, quando si riesce a fare un falso in bilancio, a quel punto si può scegliere come utilizzare questo falso in bilancio, cioè le cose che sono scappate dalle regole europee. Tremonti lo fece, per esempio, mettendo 30 miliardi di debito pubblico sulle Ferrovie dello Stato, in modo tale da nascondere quelle somme al rapporto deficit-PIL guardato dall'Europa e con quei 30 miliardi fece l'Alta Velocità Milano-Roma, un'infrastruttura che ancora adesso serve a tutti.

Il punto è che abbiamo un DEF che ci fa riflettere su cosa fare per il futuro. Teniamo presente che abbiamo sempre più vincoli mentre dobbiamo averne di meno.

a buttarlo sull'occupazione, a cercare di far sì che migliori la produttività. Questo è in parte quello che sta facendo il Governo e il fatto che ci siano 600.000 occupati in più lo indica. Ritengo pertanto che siamo nella direzione giusta, pur utilizzando delle cifre ridotte, teniamo presente per il futuro che queste cifre piccole devono diventare più grandi. Pertanto, dal mio punto di vista, attenzione: più Italia, meno Unione europea. Signora Presidente, colleghi, nell'anno che ci porta alla terza manovra di bilancio del Governo Meloni ci saremmo aspettati un Documento di economia e finanza con una prospettiva politica e un indirizzo chiari, ma ad ascoltare i colleghi dei Gruppi di maggioranza ho la sensazione che questa speranza sia vana.

un Parlamento, al quale nella seconda manovra di legislatura è stato vietato alla maggioranza di presentare gli emendamenti, avesse un sussulto di dignità davanti ad un DEF che non è un DEF, come ci ricordava il senatore Monti nel suo intervento. Ci saremmo aspettati, signora Presidente, che la si smettesse di fare opposizione all'indietro, come in una felice metafora ci ha ricordato il senatore Manca. Mai come in questo momento, per le sfide che abbiamo di fronte, avremmo avuto bisogno di condividere con la maggioranza le ricette sulla condizione del Paese. In quest'Aula - presidente Zaffini, presidente Gasparri avevate detto che gli interventi fatti l'anno scorso dal Governo sarebbero stati tramutati in strutturali con il Documento di economia e finanza di quest'anno. Non solo avete rivisto tutte le previsioni dell'anno scorso in maniera peggiorativa. Ma vorrei ricordare a tutti noi che l'anno scorso il ministro Giorgetti aveva previsto un PIL in salita, che invece ha dovuto rivedere in discesa. Vorrei ricordare che aveva previsto un *deficit* più basso, che invece avete corretto in rialzo. Vorrei ricordarvi che aveva previsto un debito più basso, che abbiamo corretto in rialzo. Questi sono i risultati che avete ottenuto con un DEF programmatico, collega Borghi. Non oso immaginare che cosa accadrà quest'anno. Veniamo al tendenziale: avete deciso di nascondere la verità al Parlamento, lo fate ininterrottamente da diciotto mesi *(Applausi)*, perché il Parlamento non è rispettato da questo Governo, perché il Parlamento è sistematicamente calpestato da questo Governo. Vorrei ricordare al ministro Giorgetti voglio ricordare soprattutto ai colleghi di maggioranza, che negli ultimi sei anni di vita di Governo ne ha trascorsi quattro anni e mezzo e, quando parlate di chi c'era ieri, chiedetevi prima che cosa vi dice il vostro Ministro dell'economia

la Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei conti, l'Istat dicono a tutti noi che non cresceremo forse nemmeno della metà, il problema non è suo: il problema è degli italiani e delle italiane *(Applausi)*. Il problema è della sanità pubblica, il problema è della scuola, il problema è di tutti quei lavoratori che lavorano. Sì, è vero che rientrano dentro la misurazione del tasso di occupazione, ma sono sotto la soglia di povertà, perché i salari non sono adeguati. Voi invece avete detto no al salario minimo. Avremmo voluto discutere, sottosegretario Freni, delle diverse terapie e delle diverse ricette. Invece, ci sono le ricette dell'opposizione, che possono essere contestate o no, ma ci sono, e non c'è alcuna ricetta della maggioranza. Non vi è consentito proporre ricette e quando ci provate, come avevate tentato con il modello Achille Lauro 4.0 l'altro giorno, tornate subito indietro perché vi rendete conto che non avete nemmeno gli strumenti per costruire misure di spesa. costruire misure di spesa. Vorrei dire una cosa molto chiara in quest'Aula, sottosegretario Freni; noi ce la siamo detta in Commissione, ma vorrei condividere con l'Aula la nostra preoccupazione. Non venga in mente alla maggioranza - lo dico al Presidente della Commissione bilancio di modificare, in nome dell'Europa, che ha modificato il ciclo di bilancio, anche la legge di contabilità, che cambiammo nel 2016 dopo due anni di indagine conoscitiva, dopo due anni di confronto tra maggioranza e opposizione di allora e approvandola con l'80 per cento del voto parlamentare, l'altro 20 si era astenuto e nessun voto contrario. Voglio ricordarlo: è stata approvata Non venga in mente a nessuno di cambiare la legge di contabilità per consentire al Ministero dell'economia di avere mani libere sulla spesa durante l'anno, per spostare risorse da un'amministrazione all'altra, perché sarebbe l'ultimo atto eversivo di un Governo che non rispetta le regole. Ve lo diciamo oggi, perché i *rumor* sull'impossibilità di fare le cose perché non ci sono mani libere aumentano e si sommano ad un attacco vergognoso del Governo ad un tempio, ad un tempio, che non dovrebbe mai essere profanato, ovviamente laico, che è la Ragioneria generale dello Stato. Non vi permettete di mettere le mani sulla Ragioneria generale dello Stato. Gli alti funzionari dello Stato non hanno una maglietta politica, non appartengono né alla destra né alla sinistra. È diventato lo sport di moda per il Governo, non potendo scaricare la colpa sul Parlamento, dire che le cose non si possono fare perché ci sono dei burocrati nascosti,

secondo semestre, in tutto il 2023 e nel primo semestre del 2024 c'eravate voi. La legge dell'agosto scorso porta la firma di Giorgetti e Meloni *(Applausi)* e consente alle villette unifamiliari di avere il superbonus pieno. Potevate fermarla. Lo avete fatto? No. Assumetevene la responsabilità fino in fondo. Veniamo alle procedure di infrazione, che vi appassionano tanto. Quando siete venuti in quest'Aula, ci avevate detto che la proposta iniziale del commissario Gentiloni non era adeguata e che avreste negoziato a Bruxelles condizioni migliorative. Io spero che il consulente non sia stato il senatore Claudio Borghi. Se il consulente è stato il senatore Borghi, allora, dal suo punto di vista, queste sono condizioni migliorative. Io penso che mai, nella sua vita, egli avrebbe immaginato che il suo sogno di avere un DEF senza numeri tendenziali sarebbe stato realizzato. Siete riusciti a farlo: il problema è che state facendo un disastro per il Paese. Quando ci avete detto che avreste negoziato, abbiamo detto di non essere d'accordo, che lo contestavamo, ma di voler vedere dove sareste arrivati. Vorrei ricordarvi che siete arrivati nella condizione in cui, in nome del MES spostato, avete svenduto l'Italia ad un negoziato, che, inevitabilmente, è peggiorativo rispetto alla prima proposta del commissario Gentiloni, ma che ci obbliga, con grande senso di responsabilità, a dire con chiarezza che non siete affidabili. L'impegno che avevate assunto lo avete smentito anche davanti al Parlamento europeo. Qualcuno dirà: ma vi siete astenuti anche voi. È vero: ci siamo astenuti, perché eravamo e siamo convinti che la proposta del Commissario agli affari economici fosse la stella polare dalla quale ripartire. Voglio aggiungere una cosa per i colleghi dell'opposizione

i tedeschi di un partito politico di estrema destra, AFD; lo hanno dato i fiamminghi del Belgio, che rivendicano l'indipendenza, lottano contro l'immigrazione e sono antiabortisti e contro le unioni omosessuali; lo hanno dato l'FPO austriaco, partito filo-Putin. State attenti, colleghi dell'opposizione, perché utilizzando la scorciatoia della propaganda non si costruisce un'Europa migliore. Ve lo dico ricordandovi che cinque anni fa insieme abbiamo lavorato per far passare alcuni di voi dai cortei dei *gilet* gialli a votare David Sassoli e vogliamo ritornare lì l'anno prossimo, a costruire un'Europa comunitaria, un'Europa che smentisce la destra oggi al Governo; un'Europa che mette insieme la difesa, che mette insieme i salari e il *welfare*; che mette insieme, oltre alla bandiera ed alla moneta, i sogni dei popoli europei. È questa la scommessa che ci giocheremo tutti alle prossime elezioni europee. Non si nasconda, senatore Borghi, con il partito più più a destra di questo Emiciclo. Dovreste invertirvi, perché sono evidenti le posizioni che state assumendo in Europa e anche il voto dato in Europa. signor Presidente, siamo consapevoli che siamo entrati in un rettilineo molto pericoloso, che sarà condizionato dalla modifica delle regole connesse al ciclo del bilancio in Europa che toccheranno le modifiche della legge di bilancio alla quale vogliamo partecipare. Abbiamo il diritto di dire la nostra e abbiamo il diritto anche di votare a favore, perché quelle regole garantiscono la Repubblica e la contabilità della Repubblica. Quello che non possiamo consentirvi è che le bugie...

colleghi, ha concluso il suo intervento dicendo che il debito costa e che questo costo sottrae risorse a cose più importanti, come sanità e istruzione. Colleghi della maggioranza, non si chiamano cose sono diritti universali e non vi permetteremo di cancellarli.

il mio saluto e la mia solidarietà alla collega Ester Mieli *(Applausi)* per l'attacco ricevuto: questa mattina, durante un'intervista alla radio, un giornalista si è permesso di eccepire sulle origini culturali e religiose della nostra collega. Spesso succede che chi si imbatte in una donna non ne esca bene e ne esca malconcio, ma guai a sfidare una donna di Fratelli d'Italia. Quindi, grazie Ester *(Applausi)* per la capacità che hai avuto di saper rispondere. Andando a parlare del DEF, vorrei in particolar modo rispondere alle accuse, che ormai sono diventate petulanti e che hanno contraddistinto audizioni, articoli di giornale ed interventi, sul fatto che il quadro tendenziale non sia programmatico. Per definizione, un quadro tendenziale non è un quadro programmatico. Le motivazioni sono state espresse e ripetute più volte, ma dovrebbe bastare il fatto che si stanno riscrivendo le regole della contabilità dell'Europa. Quindi, sarebbe ridicolo oggi applicare delle regole vecchie a un sistema nuovo che si va rinnovando. Il piano fiscale e strutturale di medio termine, che vede la scadenza del 20 settembre, farà luce su tutto quello che avete chiesto in quest'Aula e che avrà le giuste risposte. ci sarà una nuova Europa dopo l'8 e il 9 giugno e quella nuova Europa scriverà delle regole *(Applausi)* che sono nettamente meno penalizzanti nei confronti della Nazione Italia; quelle regole penalizzanti che vi hanno visto nel tempo abbassare costantemente la testa.

di propaganda, quella che ormai avete acquisito come *modus operandi* dopo che avete nel tempo condizionato pesantemente l'economia non soltanto con i vostri Governi, ma anche con quelli che sono seguiti.

gioia rispetto ai risultati ottenuti, a coloro ormai che prendono le distanze rispetto a una misura che non vogliono più sentire appioppata nei loro confronti e avvicinata ad alcune bandierine partitiche; fino alla critica del presidente Monti. Presidente, si rende conto cosa accade quando si dà ragione al centrodestra o quando non si attacca il centrodestra? Si viene criticati e quindi è toccato anche a lei.

parlamentare di bilancio affermano alcune verità sul superbonus, certamente non possiamo più omettere di aprire una riflessione da questo punto di vista. E ve lo dice chi non è stato mai uno strenuo oppositore dell'idea del superbonus, ma dell'applicazione sì, perché le misure *shock* esistono, in particolar modo nei momenti di difficoltà economica. Ma prevedere delle misure a debito senza un tetto di spesa, così come è stato fatto con il superbonus, è criminale. *(Applausi)*. È questo che stiamo pagando che continueremo a pagare per i prossimi anni; tant'è vero che, quando finirà l'effetto del superbonus, verranno fuori i dati reali di un'economia che porta a un ribasso del debito pubblico e del *deficit*. È finito il tempo del tutto gratis, è finito il tempo dell'assistenzialismo, è finito il tempo del reddito di cittadinanza, è finito il tempo della costruzione e ricostruzione gratuita su tutto. Ormai il libro dei sogni non c'è più: c'è un Governo che parla chiaro, che parla chiaro all'Europa e assume un livello di responsabilità che sta dando credibilità a tutti noi, a tutta quella Nazione che oggi aspetta un sussulto di orgoglio da parte di un Esecutivo che deve riscattare l'immagine negativa di un Paese che nel tempo non ha brillato in credibilità. Si parlava prima di una nuvola - come diceva il sottosegretario Freni - difficoltà che hanno costellato e stanno costellando il nostro percorso: due guerre, il superbonus, il Patto di stabilità, la nuova regola di contabilità che l'Europa ci chiede. Noi abbiamo incontrato queste tempeste lungo il nostro percorso, ma Darwin diceva chiaro che è destinato a vincere non chi è più forte o più intelligente, ma chi ha la capacità di adeguarsi al cambiamento. Ebbene, noi abbiamo avuto e stiamo avendo la capacità di adeguarci a tutto quello che di negativo avete combinato voi e che sta succedendo nel mondo. Oggi c'è un Governo responsabile. Mi avvio alla conclusione, caro Presidente. Noi non siamo quelli che si lamentano del vento,

che detti delle regole meno penalizzanti per il sistema Italia. Gli italiani lo stanno capendo, lo hanno capito e continuano a darci fiducia. Lo hanno fatto in Regione Abruzzo e lo hanno fatto in Basilicata, con il rinnovo del Governo di centrodestra. *(Applausi)*. Permettetemi un saluto e un ringraziamento al collega Rosa per la grande attività svolta. *(Applausi)*. Riconoscendo il lavoro svolto dal MEF, dal Sottosegretario, dagli uffici e da tutti coloro che si stanno barcamenando in questo momento di difficoltà e auspicando che con Giorgia Meloni l'8 e il 9 giugno in Europa andremo a scrivere regole nuove a beneficio di un territorio nazionale che non merita più di essere mortificato

mio intervento esprimere apprezzamento per la decisione del sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, che con lungimiranza ha colto una grande occasione per rimediare a una polemica insorta attorno alla statua cosiddetta della donna che allatta. Si tratta di una statua che

Grazie. Si tratta di una statua che tiene tra le proprie braccia un neonato e si pone nel gesto di allattare questo bambino. Il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, insieme al Senato della Repubblica, che pare proprio il giorno 6 maggio, ospiterà questa realizzazione artistica, si pone nella scia di coloro che invece hanno deciso di riconoscere il segno della maternità in essa, senza rifiutare che questa visualizzazione della madre che allatta un bambino possa andare incontro alle critiche di qualcuno. come nella storia dell'arte, dell'immagine della maternità, che in qualche modo è impressa anche in opere artistiche di altissimo livello. Non si comprende quindi come possa essere nata questa polemica milanese, forse frutto dell'idea di qualche esperto che ha preso una improvvida decisione, mettendo in difficoltà anche l'amministrazione comunale.

È stato un prete intransigente sui princìpi, disponibile al dialogo a tutto campo, magnanimo e misericordioso con i più deboli, ma è stato anche un giornalista con la schiena dritta e con la penna felice alla perenne ricerca della verità, - come diceva - ogni medaglia ha il suo rovescio e spesso ciò che sta dietro è più di quello che si vuol far vedere e credere. Nato nel 1930, il 28 novembre, per più di vent'anni è stato il direttore del settimanale diocesano «Vita Trentina», presso il quale ha allevato una pattuglia di giornalisti che poi hanno frequentato altre chiese, sono approdati in altre parrocchie, dalla RAI all'Ansa, all'AGI, all'Alto Adige e all'ufficio stampa della Provincia, senza mai dimenticare le origini e gli insegnamenti del maestro. Vittorio Cristelli ha varcato la soglia dell'infinito dopo una vita intensamente vissuta. Ha studiato filosofia all'Università di Padova, dove si è laureato nel 1965. Dal 1967 al 1989 è stato direttore del settimanale diocesano «Vita Trentina», mentre dal 1962 al 2005 ha svolto l'attività di docente alla Scuola di servizio sociale. È stato consigliere nazionale dell'ordine dei giornalisti e vice presidente del sindacato dei giornalisti. Considerato una delle penne più brillanti del giornalismo trentino, don Cristelli ha sempre rivendicato quale caratteristica del giornalista il ruolo di cane da guardia nei confronti del potere politico, economico e sociale e il giornalismo come voce di chi non ha voce. Ringrazio Alberto Folgheraiter, suo allievo, per il prezioso contributo a questo intervento di ricordo.

È l'ennesima condanna del regime iraniano di ragazze e ragazzi che partecipano alla protesta nota anche da noi come «Donna, vita, libertà». Qual è la colpa di Toomaj? Aver scritto le parole di una canzone dopo l'assassinio di Mahsa Amini, nota come la ragazza che ha dato vita - e dato il via, anche - al grande movimento di liberazione delle donne iraniane. Si parla poco della lotta delle donne iraniane, che continua dentro una repressione sempre più feroce. Il coinvolgimento della Repubblica dell'Iran nel conflitto mediorientale in realtà è stato l'alibi attraverso il quale il Governo ha dato una stretta alle misure di repressione del suo popolo e delle sue donne.

Per questo, signor Presidente, tramite lei, vorrei chiedere al Governo innanzi tutto di fare una protesta effettiva per impedire che questa ennesima condanna si realizzi e che quindi il giovane Toomaj possa continuare a vivere *(Applausi)* e per continuare

quante vite valgono alcuni rapporti commerciali o magari i rapporti che ci sono tra Paesi. Ci dev'essere un momento in cui proviamo a dire che prima vengono i diritti e le libertà delle donne e dei ragazzi e poi gli altri interessi. Per questo credo sia giusto chiedere al Governo di manifestare